di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria

Signora Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 2165, che l'Assemblea si accinge ad esaminare, è stato, come noto, già approvato dalla Camera dei deputati e oggetto, nel corso della scorsa settimana e della giornata passata, di un proficuo dibattito presso le Commissioni riunite 6a e 10a del Senato. L'attenzione riguardo a questo documento e alla sua definizione è molto alta, perché introduce misure che reputo di vitale importanza per l'economia del nostro Paese soprattutto in questa fase delicata: disposizioni - come recita il titolo del disegno di legge - per il contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, potenziamento e razionalizzazione...

signora Presidente. Potenziamento, dicevo, e razionalizzazione della riscossione tributaria che ci consente di adeguarci alla normativa comunitaria e

questi incentivi hanno permesso di aprire circa 350.000 domande, quindi ci sono già 350.000 richiedenti sui beni oggetto di questi incentivi. Addirittura il presidente del CECED, che è uno degli organismi di Confindustria che si occupa in maniera specifica di questi beni, che dichiara l'alta rispondenza di questo dispositivo alle attese dell'industria nazionale. imprenditoriale - destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Si tratta di un atto molto articolato e organico nel perseguire un obiettivo che sta a cuore a chiunque creda nel nostro sistema Paese: un sistema che in passato ha dimostrato grande forza, di cui oggi ancora conserva saldamente le potenzialità, che ritroviamo nel patrimonio di competenza e di intraprendenza a cui il decreto di cui stiamo discutendo vuole offrire strumenti di sostegno e stimolo. Il momento è sicuramente molto complesso: la crisi greca ci ha messo di fronte ai rischi di politiche dissennate nel permettere stili di vita al di sopra dei propri mezzi. L'Italia ha giocato un ruolo determinante nel salvataggio della Grecia. L'azione del presidente del Consiglio Berlusconi, coordinata con quella dei Capi di Governo delle maggiori potenze europee, ha dato buone garanzie di stabilità finanziaria all'Unione. E su questo mi permetto di agganciarmi a quanto sta avvenendo nel settore della moneta unica, quindi al rapporto euro-dollaro. Negli ultimi giorni si parla di un euro debole. Ebbene, mi sento di affermare che euro debole significa industria italiana forte.

Nella mia esperienza imprenditoriale già sento commenti da parte di imprenditori nazionali che vedono i competitori cinesi alzare i propri listini nel mercato europeo. Sta diminuendo quindi il *gap* competitivo che il nostro Paese ha sempre avuto nei mercati internazionali, e in questo momento la nostra posizione si sta rafforzando grazie all'azione del nostro Governo verso la finanza internazionale e grazie al fatto che l'euro non si sta indebolendo ma sta tornando ai valori di giusto peso rispetto alla moneta internazionale. Se in questa circostanza abbiamo potuto giocare da protagonisti è anche grazie alla credibilità che il nostro Governo ha conquistato nel corso della crisi globale con cui abbiamo dovuto fare i conti nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo sofferto e soffriamo, ma la nostra tenuta è un dato di fatto. La nostra politica economica e finanziaria ci ha presentato come Paese virtuoso nelle compagini europee, e questo lo dobbiamo alle misure severe adottate dal Governo Berlusconi e, nella fattispecie, dal ministro Tremonti. In questi frangenti sono indispensabili azioni di responsabilità, regole e provvedimenti improntati al rigore e all'oculatezza e, ne sono certo, questo disegno di legge offre un importante contributo in questa direzione. Un esempio di questa mattina è l'aumento della produzione dell'acciaio inossidabile. L'economia mondiale sta tornando a correre, e con essa anche l'Italia. Rispetto a quanto dicevo poc'anzi sulla valuta e sul vantaggio competitivo dell'Italia, abbiamo l'informazione che la produzione dell'acciaio inossidabile è cresciuta del 59 per cento: è un dato che non si registrava da un trentennio. Ci ritroviamo, anno su anno, con un aumento di circa il 60 per cento della produzione di acciaio inossidabile mondiale. Ricordo che l'acciaio inossidabile è uno dei principali componenti nella costruzione

Mi soffermerò più avanti su questo aspetto, anticipando però che riconosciamo che il capitolo spesa è contenuto ma, allo stesso tempo, stesso tempo, sufficiente per una serie di interventi non solo efficaci, ma anche salutari per l'iniezione di fiducia che sapranno imprimere all'economia, alle imprese e al mondo del lavoro,

che in Europa la crisi si sente, ma è altrettanto vero che in molti Paesi emergenti, come Cina, India o Brasile l'economia ha ripreso a correre. Sulla Cina e l'India

che tale sistema non può diventare un peso: anzi, dobbiamo fare in modo che queste dinamiche internazionali siano sempre al centro del nostro ragionamento.

sono queste ultime che possono fungere da volano per un'economia come quella italiana, dove la vocazione imprenditoriale è forte e dove sono ancora numerosi i casi di eccellenza

all'allora ministro Bersani, il quale ci spiegava la politica industriale del precedente Governo. Ebbene, io mi permisi di svolgere un intervento richiamando la passione richiamando la passione dell'intraprendere verso la passione della politica; ricevetti, però, dall'allora ministro Bersani

a trasmettere la passione di intraprendere ai nostri imprenditori, che ci hanno portato fin qui, che hanno dato alla nostra Nazione quello slancio che oggi ci permette di affrontare la crisi a testa alta, di guardare negli occhi il dramma che sta vivendo la Grecia e poter giocare da protagonisti nell'azione di salvataggio, non della Grecia, ma di tutto il continente europeo. Ora, quindi, serve uno scatto di orgoglio da parte di chi fa impresa, un cambio di passo che consenta di adeguare le capacità dei nostri imprenditori a ciò che il mercato chiede, sfruttando al meglio le opportunità che esso ci offre. Essere in un mondo che cambia non vuol dire regredire: anzi, per chi ha una disposizione naturale al cambiamento, come chi fa impresa e come dovrebbe avere chi fa politica, questo è il momento di mettersi in gioco. Non si cresce se si resta uguali a se stessi, e le rotture sono i frangenti in cui possiamo metterci in discussione ed evolvere. Fino a ieri, non più di quindici anni fa, era impensabile per un imprenditore italiano dover competere con un imprenditore cinese o indiano, come era improbabile che un imprenditore italiano dovesse poter apprendere come fare impresa o realizzare prodotti da un cinese o da un indiano. Oggi questa è la normalità con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente, con molto realismo; umiltà, ma senza perdere lo spirito che è alla base di chi vuol fare impresa: la voglia di fare, di rinnovarsi ogni giorno, di cercare buone idee. Questa premessa è indispensabile per cogliere a fondo il senso del disegno di legge che andremo a discutere: le misure che introduce sono strumenti che possono sostenere gli imprenditori nella loro attività, ma non possono sostituirsi a quel presupposto imprescindibile per un imprenditore che è la capacità e la voglia continua di giocare la propria carta vincente, mettendosi in discussione, se necessario. Se è vero che le risorse riferite a questo decreto sono contenute, è altrettanto vero che le misure sono valide. È un atto fortemente coerente con le sue finalità e con il contesto da cui è scaturito. Utilità, serietà e rigore potrebbero virtualmente essere i tre assi portanti di questo disegno di legge. Un segnale forte di serietà e di rigore è senza dubbio il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, lotta che sarà una

che si realizza attraverso lo specifico sistema dei «caroselli» e «cartiere», un circuito commerciale tra imprese operanti nell'Unione europea, al cui interno si provocano solo formalmente dei movimenti a catena, grazie alla presenza di società «cartiere» (che producono solo carta, vale a dire fatture) e di società filtro. Le somme recuperate riversate allo Stato restano quindi acquisite all'erario. In merito al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nel quale si prevedono disposizioni volte a garantire il «rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali», si rileva l'opportunità di specificare adeguatamente a quale tipologia di concessioni pubbliche si fa riferimento, tenuto conto che le disposizioni del comma 2 e dei commi successivi riguardano specificatamente il settore dei giochi. La genericità della definizione del soggetto destinatario della norma non corrisponde, infatti, alla disciplina ad esso indirizzata, che ha la finalità di intervenire sul settore dei giochi. La necessità di chiarire la definizione di «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali» è stata peraltro segnalata dalla relazione al testo del decreto-legge del Servizio studi della Camera dei deputati. Alla luce di quanto sopra esposto, si suggerisce quindi di delimitare la tipologia di concessione pubblica statale, come relativa al settore dei giochi, anche al primo periodo del comma 2. Nel testo, inoltre, è previsto l'adeguamento alla direttiva Ecofin in materia di notifiche ai contribuenti non residenti in Italia: esse si considerano validamente effettuate con la spedizione della raccomandata (con avviso di ricevimento) all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. La notifica ai contribuenti non residenti è poi validamente effettuata, qualora i medesimi non abbiano comunicato al fisco l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti. Le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente anche ai fini della riscossione. Siamo quindi di fronte ad un provvedimento di modernizzazione e di trasparenza che non potrà che migliorare e rendere più responsabile il rapporto tra cittadini e Stato. Al l'introduzione della posta elettronica certificata: un altro degli obiettivi raggiunti dal nostro Governo, e che quindi riteniamo possa ricollegarsi a questa parte del disegno di legge Sul piano delle liberalizzazioni, credo sia giusto soffermarsi anche sull'articolo 5, per le attività di edilizia libera: un rilancio del piano casa, che consentirà di effettuare lavori interni, a meno che non ci sia una legge regionale che lo vieti.

anche per via telematica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori. Il provvedimento d'urgenza, che il Governo ha deciso di adottare verso la fine di marzo, era stato più volte richiesto da diversi settori destinatari degli incentivi, al fine di assicurare, in un momento di crisi economica di carattere internazionale, un adeguato sostegno alla domanda. Come ho avuto modo di sottolineare anche nel corso dei lavori delle Commissioni riunite, il provvedimento varato dal Governo costituisce un intervento particolarmente coraggioso in una fase come quella attuale. Ricordo infatti che diversi Paesi europei nelle ultime settimane, a seguito dell'esplosione della crisi greca, hanno dovuto varare politiche assai rigorose per un contenimento complessivo della spesa pubblica. italiano, nella consapevolezza che gli interventi già promossi negli ultimi mesi stanno consentendo all'Italia, anche secondo le stime recenti del Fondo monetario internazionale, di affrontare con maggiore serenità*...

il decreto-legge in esame, approvato il 6 maggio scorso dalla Camera dei deputati e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato significativamente ampliato in prima lettura con una serie di misure che concernono molti degli ambiti già presenti nel testo originario, con particolare riguardo ai seguenti profili: contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, potenziamento dell'amministrazione finanziaria, razionalizzazione della riscossione, misure sui giochi e interventi agevolativi a sostegno della domanda. Sulle disposizioni concernenti gli incentivi ha ampiamente riferito il senatore Casoli. Per quanto mi riguarda, chiedo alla Presidenza di poter consegnare una relazione illustrativa delle misure di competenza della 6a Commissione. Tre soli accenni, o sottolineature, nel merito: le misure sui giochi tendono a consolidare l'indirizzo di garantire maggiore legalità, trasparenza ed efficacia dei controlli, nonché a garantire il mantenimento del gettito erariale; le norme in materia di riscossione tendono a risolvere alcune complesse e non più rinviabili questioni; infine, la Camera dei deputati ha inserito una disposizione sulla devoluzione del 5 per mille, rifinanziando anche l'anno 2011. Senza sminuire il testo approvato, avremmo certamente preferito far proseguire l'*iter* dei disegni di legge in tale materia già avviato dalla 6a Commissione. Come dicevo, onorevole Presidente, il senatore Casoli è ampiamente intervenuto sul merito del provvedimento. Ritenendo di non travalicare il mio ruolo di relatore nella misura in cui mi ricollego comunque ad un lungo e approfondito confronto avviato nella Commissione finanze, non intendo sottrarmi al compito di esprimere una pur sintetica valutazione politica sul decreto in esame. Esso è frutto di una congiuntura che, maturata pochi mesi fa, appare già - direi purtroppo - ampiamente superata: un provvedimento che unisce misure del gettito erariale e di redistribuzione di incentivi ad alcuni settori produttivi non sembra oggi strada né esaustiva, né ottimale. Infatti, da un lato, le condizioni della finanza pubblica appaiono tali da suggerire cautela e prudenza nella gestione dei capitoli di spesa più problematici, dall'altro, la scelta di incentivare alcuni settori produttivi mostra evidenti limiti sia strategici che finanziari. Come più volte emerso da dibattiti all'interno della nostra 6a Commissione, appare a molti potenzialmente più efficace concentrare le misure sui fattori produttivi e non su singoli settori. Occorre guardare ai prossimi appuntamenti leggendo le dinamiche della crisi e gli scenari che si aprono con un po' più di attenzione: il ministro Tremonti, nella predisposizione delle linee d'intervento per il prossimo biennio, e il Governo, nelle scelte che si appresta a compiere, sono certamente e fortemente consapevoli della necessità di una mirata incisività soprattutto sul fronte delle spese. Come ho già avuto occasione di accennare ieri nei lavori delle Commissioni riunite, auspico che maggioranza e opposizione - magari partendo qui, dal Senato - sappiano creare l'occasione per fornire elementi costruttivi di confronto sulle linee d'intervento sulle quali si dovranno presto misurare Governo e Parlamento. Nessuno può pretendere di avere una risposta risolutiva, ma tutti abbiamo consapevolezza che scelte di rigore sulla finanza pubblica evocano una condivisione che deve essere il frutto di una profonda e concreta responsabilità istituzionale.

*Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, in premessa vorrei sottolineare che per l'ennesima volta discutiamo di un provvedimento di misure fiscali e di sostegno all'economia in quest'Aula compiendo sostanzialmente una finzione, perché siamo a ridosso dei termini di decadenza del provvedimento se non convertito e, dunque, subiamo una limitazione degli spazi di confronto e delle possibilità di modifica praticabili in questo ramo del Parlamento.* Per la verità, non c'è solo poco tempo per discutere: c'è anche molta poca materia su cui confrontarsi, posta la limitatezza e l'esiguità delle misure incentivanti e di sostegno dell'economia e per un rilancio di talune tipologie di consumi contenute in questo provvedimento. Prendo a prestito il commento icastico di una mia concittadina, la professoressa Maria Cecilia Guerra, pubblicato su «La Voce»: «Nel complesso, un decreto senza personalità, poco utile sul piano economico, con costi di attuazione da non sottovalutare», - con poche risorse: 420 milioni di euro in totale, di cui 150 rappresentano - anche questa non è una novità - un diverso utilizzo di fondi già stanziati. Il resto è finanziato con fondi che arrivano da norme antievasione ed orientate a sostenere una somma di microinterventi distribuiti su vari settori che, certo, a qualcosa serviranno, perché nella difficoltà generale che attraversiamo tutto serve, ma difficilmente solleciteranno nuova domanda. Però va riconosciuto l'effetto spot, che è poi ciò che si voleva ottenere: ebbene, c'è stato e lo si è fatto ben valere per le elezioni regionali, secondo una prassi consolidata per questa maggioranza e il suo Governo. Oggi, però, il contesto in cui valutiamo questo provvedimento costringe anche voi a fare i conti con la realtà. Discutiamo questo decreto dopo le vicende drammatiche che si sono manifestate in Grecia, la ripresa di turbolenza dei mercati finanziari, l'attacco alle economie più vulnerabili dell'eurozona e alla stessa stabilità dell'euro, nonché a seguito di decisioni assunte in ambito europeo da Governi, Commissione, Banca centrale europea e nell'imminenza di manovre di correzione dei conti che sono annunciate per tenere l'Italia al riparo da minacce speculative e allinearsi ai criteri di rigore definiti su scala europea. Insomma, non è davvero più tempo di furberie e di *escamotage*: bisogna che anche il Governo e la sua maggioranza si lascino alle spalle le stagioni della mera ed effimera propaganda per assumersi le responsabilità che il momento richiede. Ricordiamo tutti le affermazioni, risalenti solo a qualche settimana fa, del ministro Tremonti secondo le quali la crisi economica era ormai alle nostre spalle e non erano necessari ulteriori interventi di sostegno dei consumi e della produttività. La realtà dei numeri e le recenti vicende evidenziano, al contrario, che per il nostro Paese gravi problemi stanno ancora drammaticamente di fronte a noi. In questo senso, i dati della Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, confermati anche in sede europea e dalla Banca d'Italia, evidenziano una situazione assai seria in cui ci troviamo, dopo anni un po' più lontani in cui, grazie ad iniziative di contenimento della spesa pubblica, si era conseguito un costante rientro del debito pubblico verso la soglia del 100 per

il saldo primario risulta in disavanzo, la spesa corrente (al netto degli interessi) raggiunge il 43,4 per cento e la pressione fiscale si è accresciuta nel 2009 fino a raggiungere il 42,8 per cento del PIL e si manterrà vicino a questa soglia record fino al 2013, cioè per l'intera legislatura. Pertanto, mentre da un lato non si sono prodotti sforzi adeguati per frenare la caduta della ricchezza nazionale, dall'altro il tanto sbandierato rigore nella tenuta dei conti pubblici, di cui abbiamo sentito cenni anche nella relazione del relatore Casoli, è clamorosamente smentito dai numeri e dai fatti. Lo diciamo con nettezza: la gravità della situazione in cui si trova il Paese non può essere attribuita per intero e soltanto alla crisi economica e finanziaria internazionale. Molto dipende ed è dipeso dall'immobilismo del Governo in questi due anni e dalla reiterata sottovalutazione dei problemi del Paese. La dinamica di medio periodo prevista per la nostra economia è molto modesta in confronto a quella dei principali Paesi concorrenti e, soprattutto, inadeguata a fronteggiare le sfide del nuovo scenario globale e contrastare l'aumento dei disoccupati già registrato e previsto almeno fino a tutto il 2010. Anche il livello del PIL che avevamo nel 2007 sarà recuperato solo tra diversi anni. Scontiamo, quindi, una perdita di prodotto di carattere permanente, che inciderà anche pesantemente sulle problematiche di risanamento del debito pubblico. Nel frattempo, le famiglie diventano sempre più povere: il reddito lordo a loro disposizione è sceso vertiginosamente, con inevitabili ricadute sul livello generale dei consumi. Cade, poi, purtroppo incrinandosi un po' - ed è questo un segno allarmante - uno dei fattori fondamentali della nostra economia: il risparmio delle famiglie, finora sempre al di sopra del livello registrato nel resto dell'Europa e degli USA, oggi invece si attesta al livello medio europeo. In sintesi, l'analisi del quadro economico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico, ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro. Non è certo la prima volta che lo diciamo e continueremo ad incalzare la maggioranza perché si cambi approccio e si correggano gli errori compiuti. Per questo apprezziamo, ad esempio, nel provvedimento al nostro esame le misure di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie a livello internazionale, perché l'evasione e l'elusione fiscale sono uno dei pochi ambiti su cui è possibile incidere per recuperare risorse, facendo equità, rimuovendo distorsioni nel mercato, indirizzando anche quelle entrate che possono essere così raccolte particolarmente a sostegno di manovre di più equa ripartizione del carico fiscale sulla platea dei contribuenti. In questo senso, il contrasto alle frodi «carosello» è meritevole, ma è ancora una misura troppo timida; sarebbe stato molto meglio per contrastare tutte le frodi «carosello» e più in generale l'evasione dell'IVA, se questo Governo non avesse abolito subito, nell'estate del 2008, l'obbligo (tanto esecrato, ma evidentemente poi non così inutile visto che lo si recupera e rinvigorisce) di comunicare per via telematica l'elenco dei clienti fornitori relativo a tutte le transizioni, anche quelle domestiche. C'è ancora modo di correggersi anche sulla tracciabilità dei pagamenti e l'uso della moneta elettronica: i nostri emendamenti vanno in questa direzione. Vorrei però sottolineare che la strada del ravvedimento operoso

Questa volta è toccato al contenzioso tributario, con misure che possono anche risultare condivisibili per velocizzare procedure ed introitare anticipatamente le somme attese. Quel che non convince, però, è il disposto dell'articolo 3, comma 2-*bis*, che, per quanto attiene alle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione, ne consente l'estinzione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. In merito, mi limito a citare il commento, come sempre eccellente, degli uffici del Senato: «Ad una prima interpretazione della norma sembra che ci si trovi di fronte ad una sorta di sanatoria». affermando: «Tuttavia, non è escluso che gli effetti finanziari netti della norma in questione possano essere di fatto negativi». Ciò perché decideranno di aderire a questa procedura rapida di estinzione del procedimento coloro che avranno convenienza a farlo, mentre per l'erario l'entrata sarà ampiamente minore rispetto a quanto avrebbe potuto incassare con qualche ritardo, nell'ipotesi in cui il giudizio di ultimo grado si fosse chiuso con la soccombenza del contribuente. Oltre a ciò, e mi pare che sia un tema che meriterebbe più attenzione, credo si possa riscontrare qualche non secondario profilo di delicatezza su questa decisione in tema di conflitti di interesse (mi auguro che il Presidente del Consiglio fosse almeno per forma assente quando si è approvata questa norma), posto che a più riprese nei mesi scorsi e anche in questi giorni su autorevoli mezzi d'informazione si è riferito che tra i beneficiati potesse essere annoverata anche una grande impresa, la Mondadori, di cui si dice di un contenzioso con l'Agenzia delle entrate per circa 200 milioni di euro, che potrebbe rientrare nella fattispecie sopra descritta. Ho grande rispetto per questa importante azienda nazionale, che considero un protagonista primario nel campo dell'editoria e della comunicazione, ma il Governo può dirci qualcosa di più in merito? Quali altre situazioni ricorrono, se ricorrono, insieme a quella indicata? Come dobbiamo interpretare la norma, sempre stando al commento del Servizio del bilancio, che giustamente rileva: «Riguardo inoltre al fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze accerterà annualmente le maggiori entrate, ciò sembrerebbe supporre che la disposizione in esame rimarrà in vigore a regime»? È davvero così? Vi pare cosa di poco conto da inserire furtivamente in un decreto su cui si è posta e si porrà probabilmente anche qui la fiducia ? E come si può pensare, lo chiedo al Governo, di invertire una tendenza, di chiamare il Paese a uno sforzo di coesione e partecipazione alle difficoltà, come ci invitava a fare anche adesso il relatore Conti, se la lealtà fiscale, anziché premiata, viene irrisa e c'è sempre una corsia preferenziale per chi sa essere più furbo e adeguatamente ammanicato?

per cui questa misura si presenta insieme come arrogante e irridente nei confronti della pubblica opinione. Invece delle intemerate demagogiche sugli sprechi degli enti locali, sui fannulloni

Comprendiamo le esigenze di garantire un gettito all'erario, di accompagnare le evoluzioni tecnologiche, di operare per portare ad emersione un flusso finanziario che altrimenti sarebbe appannaggio dei circuiti illegali. Tuttavia, non possiamo non constatare l'affastellamento di norme che si sono succedute in questi due anni senza un vero coinvolgimento in una discussione di orizzonte strategico sulle strategie e sugli indirizzi complessivi. Non possiamo neanche non rilevare

Non solo, pensiamo si dovrebbe dedicare qualche riflessione ad alcuni numeri: nei primi quattro mesi del 2010 si è registrato un aumento delle perdite legate alla dipendenza da giochi e scommesse di In Italia, il solo gioco legalizzato coinvolge circa 29 milioni di persone e sviluppa un fatturato di circa 54 miliardi di euro; il coinvolgimento dei minorenni è aumentato, passando da 860.000 unità a quasi 2 milioni. Penso che questi dati bastino a dare il senso della necessità di una seria disamina del fenomeno

del vice presidente del senato Chiti e del presidente del Gruppo PdL Gasparri. Soprattutto, però, ci preme mettere in evidenza che il testo così come articolato alla Camera apparentemente vuole dare un sostegno al terzo settore, ma per il modo in cui è stato scritto crea le condizioni perché gli vengano sottratte risorse, penalizzandone la possibilità di ricevere sostegno ed aiuto per la preziosa opera di coesione sociale e per la costruzione di un senso di comunità solidale di cui il volontariato ed il settore *no profit* sono una risorsa imprescindibile e fondamentale. Per quanto riguarda più analiticamente le misure le misure del Fondo per il sostegno alla domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica e quant'altro (gli interventi che si rivolgono a 10 settori e 19 tipologie di beni),

lo ha spiegato benissimo il presidente Baldassarri intervenendo nel dibattito in Commissione - la congerie di microinterventi indirizzati ai diversi settori, che in molti casi, più che sollecitare nuova domanda, inducono ad anticipazioni di spesa comunque programmate. Per economia di ragionamento e compatibilità di tempi non mi soffermo su aspetti che sono stati positivamente corretti e almeno parzialmente migliorati nella discussione alla Camera, con riferimento sia alle polizze assicurative vita dormienti che alla delicata questione della riscossione riguardante le vicende di Tributi Italia.

dibattito anche le proposte di emendamento. Anche sulla questione delle agevolazioni edilizie penso che è sempre bene semplificare la burocrazia, ma bisogna stare attenti a non produrre norme che in realtà rischiano di determinare, soprattutto

dovemmo anche noi misurarci con la "traforite" che andava di moda nell'allora Governo Berlusconi, quando alle Infrastrutture il ministro era Lunardi, molto appassionato di gallerie e di trafori. Pensare ad una metro di quel tipo era sbagliato: per dimensione, bacino di utenza potenziale, costi di realizzazione e gestione. Fummo spinti anche noi a ragionarci, perché altrimenti pareva chiamarsi fuori da chissà quale epocale occasione. Ora vedo che si torna indietro, ed è un esito in qualche modo annunciato, ma si lasciano per strada un po' dei soldi su cui a suo tempo lo Stato si era impegnato e si disperdono le risorse residue in più rivoli. Una compensazione che magari dà un po' di respiro finanziario al Comune di Parma, ma taglia fuori del tutto la Regione (che pure in precedenza era stata responsabilmente al tavolo dell'intesa di programma) e, soprattutto, mette a rischio la soluzione di problemi di mobilità rispetto ai quali progetti di minore impatto e minore costo possono costituire non solo una risposta per la città di Parma e per i suoi cittadini e le loro esigenze, ma anche una interessante sperimentazione per una più vasta platea di città medie. Insomma, anche questo piccolo esempio è la conferma di un modo di procedere confusionario, davvero molto poco federalista: ci si arrangia nell'ottica del piccolo cabotaggio, con un occhio magari alle contiguità politiche, ma così, rispetto ai problemi che vive il Paese, non si va da nessuna parte. C'è bisogno di regole, trasparenza, linearità e chiarezza di indirizzi e obiettivi. Questo provvedimento, invece, non definisce alcun obiettivo strategico - né per il prossimo anno, né per quelli successivi - sul terreno della ripresa economica; non è prevista alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese attraverso un netto accrescimento della produttività totale dei fattori. Come già ampiamente emerso nel corso degli ultimi due anni, la nostra visione dei problemi e delle modalità per affrontarli è diametralmente opposta a quella finora sostenuta dall'Esecutivo e dalla sua maggioranza ed è incentrata su un chiaro indirizzo di sviluppo per una crescita sostenibile, insieme alla necessità di correggere le crescenti, insopportabili diseguaglianze che si stanno radicando nel Paese. Nell'attuale fase congiunturale, l'Italia ha certamente problemi, ma anche le risorse sufficienti per resistere alla crisi e riproporsi da protagonista nel contesto internazionale e nel ciclo di sviluppo che verrà dopo la crisi: il nostro apparato produttivo, specie nella sua componente manifatturiera, è in grado, dopo la ristrutturazione che ha saputo interpretare, di approfittare di una possibile ripresa dei consumi nell'economia internazionale e della domanda di qualità propria del *made in Italy*, che può giovarsi dell'esistenza di nuovi consumatori apparsi di recente sullo scenario internazionale. Ma queste potenzialità - concludo, Presidente - sono destinate a restare tali; anzi, rischiano di essere mortificate e di isterilirsi se non viene in campo un progetto consapevole della politica che riduca i fattori di debolezza ed esalti quelli di forza, e soprattutto se non si abbandonano posizioni di fatto conservatrici che si oppongono, sulla base di logiche di tutele neocorporative delle situazioni di fatto e delle condizioni di rendita, all'apertura dei mercati, alla concorrenza e alle necessarie riforme strutturali del settore pubblico e privato, in un'ottica, naturalmente per noi, di equità sociale. A questi temi non potrà sottrarsi qualunque discussione sulle manovre di correzione dei conti pubblici di cui si sta ragionando in questi giorni e che probabilmente verranno portate, immagino già dalla prossima settimana, all'attenzione dell'Assemblea. Noi pretendiamo finalmente che si apra su questo un confronto serio, costruito su elementi di verità, per dare al Paese risposte che siano davvero all'altezza della sua crisi.

*(PD)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, arriva in Senato, dopo l'ennesimo voto di fiducia alla Camera, un decreto da convertire in legge che ha tra gli obiettivi di maggior rilievo quello di sostenere la domanda interna. intento certamente condivisibile in un momento come l'attuale, in cui la crisi economica e produttiva non è finita e vi è assoluta necessità di rilanciare la crescita del nostro prodotto interno lordo. Ma gli obiettivi che esso si pone sono troppo ambiziosi, purtroppo, rispetto allo strumento messo in campo: un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori,

preoccupati per l'attuale situazione di crisi, che è la più grave dal 1945. Ricordiamoci che il 2009 si è concluso con una contrazione del 5 per cento del PIL, la pressione fiscale ha raggiunto livelli altissimi (43,2 per cento), il tasso di disoccupazione è in costante aumento (i dati ISTAT di marzo registrano l'8,8 Com'è stato detto, le famiglie italiane si stanno impoverendo. Sempre dai dati ISTAT del 2009 si rileva che il reddito disponibile è diminuito del 2,8 per cento rispetto al 2008, con una grave ripercussione sui consumi. Aumentano le tariffe nei servizi regolamentati, trasporto ferroviario, servizi postali, assicurazioni auto, pedaggi autostradali: sono vere e proprie tasse occulte e nulla si fa per contrastarne la crescita. È evidente, quindi, che devono essere messe in campo misure adeguate e serie dal lato della domanda, non certo come quelle introdotte con il decreto che oggi esaminiamo. È arrivato il momento di intervenire concretamente sull'attuale distribuzione dei redditi, attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, certo per rafforzare il potere d'acquisto e incrementare la domanda interna, ma soprattutto per costruire nel nostro Paese una maggiore equità sociale. Siamo in un Paese in cui la distribuzione del reddito peggiora sempre di più, come ho detto, collocandoci tra i primi tra i Paesi OCSE per indice di disuguaglianza. Devono anche essere adottate misure di medio-lungo periodo (quelle riforme strutturali di cui in questi giorni il Governo di centrodestra parla molto, senza avere però formulato proposte concrete) che devono servire al Paese per recuperare quel *gap* che già prima della crisi ci allontanava dagli altri Paesi europei nella crescita. Un capitolo fondamentale di intervento è costituito dal supporto al sistema delle piccole e medie imprese, che sono il motore dello sviluppo economico del nostro Paese. Lo stanno dimostrano in questa situazione di crisi: cercano in tutti i modi di salvaguardare il capitale umano, riducono i costi e limano i profitti. Iniziamo ad affrontare seriamente i problemi di queste imprese, come l'accesso al credito, con la consapevolezza che si presta a chi già il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, una fiscalità più equa, la semplificazione amministrativa. Tra le politiche da affrontare per le PMI è sicuro che occorre investire di più in ricerca ed innovazione. Le imprese vanno incentivate in questo senso. La crescita della produttività in Italia è un problema, non solo perché cresce poco il PIL, ma anche perché se cresce l'occupazione ciò avviene senza che ci sia innovazione. Tra le tante contraddizioni di questo decreto c'è anche il fatto che il Fondo per il sostegno alla domanda è finanziato per 50 milioni di euro mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per spese per attività di ricerca e innovazione tecnologica. Si continua a tagliare in questo senso in attesa di fantomatici interventi ancora annunciati e non attuati. Le imprese tutte e non solo le PMI aspettano una politica industriale di medio-lungo periodo che preveda tra le altre misure quelle che facilitino le spese in ricerca e innovazione (come la defiscalizzazione degli investimenti fatti in tal senso). Quindi il Fondo per il cosiddetto sostegno della domanda è finanziato solo in parte da nuove risorse, mentre per il resto, oltre ad incidere sul credito d'imposta per ricerca e innovazione si va ad incidere sul Fondo per la finanza d'impresa. In sostanza, si finanzia la domanda con risorse destinate alle imprese per interventi di carattere strutturale. Onorevoli colleghi, a questo punto, per il tempo restante che mi è concesso, voglio trattare la vicenda delle cosiddette polizze dormienti, disastrosa per tanti risparmiatori, che a loro insaputa sono stati assoggettati ad un vero e proprio scippo legalizzato. II decreto in esame fa un passo in avanti con la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 4, ma ancora c'è molto da fare perché nessun risparmiatore perda un euro a causa di un errore commesso da questo Governo. brevemente di riassumere l'accaduto. La legge finanziaria n. 266 del 2005 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime delle frodi finanziarie: tale fondo si alimenta con le risorse dei conti correnti dormienti. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 ha regolamentato il funzionamento del fondo e ha specificato quali sono i rapporti contrattuali interessati ed i criteri per l'individuazione. In breve, si può affermare che sulla base di queste e di altre disposizioni le somme dovute ai beneficiari di polizze vita sarebbero confluite nel fondo per le vittime delle frodi finanziarie solo decorso il decennio, a prescindere dalla prescrizione del diritto. Le compagnie di assicurazione potevano rinunciare ad avvalersi del termine di prescrizione di un anno corrispondendo le somme maturate dai beneficiari di polizze vita che non le avessero richieste entro l'anno dal decesso del titolare. decreto Alitalia la situazione è cambiata e questo Governo ha previsto che nel fondo dovevano confluire gli importi dovuti ai beneficiari di polizze vita non reclamati nel termine di prescrizione. Contestualmente è stato elevato a due anni il termine di prescrizione del diritto. prevista inoltre un'applicazione retroattiva anche alle polizze per le quali gli eventi che determinano la prescrizione si siano verificati prima del 1° gennaio 2006, quando ancora si applicava la finanziaria del 2005. Gli effetti di queste norme sono stati vari. In primo luogo, a causa della retroattività della legge n. 166 del 2008 gli eredi dei titolari di polizze deceduti tra il 2005 e il 2008 hanno visto svanire senza alcun avvertimento i risparmi di una vita nel momento in cui la legge è entrata in vigore. A quest'ultima situazione si cerca di ovviare eliminando la retroattività con la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 4, ma questa previsione è insufficiente a portare chiarezza sulla vicenda perché gli importi derivanti da polizze prescritte già devoluti al fondo non possono più essere richiesti dai beneficiari. Un'ingiustizia cui occorre porre rimedio al più presto restituendo fino all'ultimo centesimo. Occorre trovare le risorse che sono state impegnate nel bilancio dello Stato distraendole ai cittadini inconsapevoli. I nostri emendamenti sono pertanto volti a rimediare a questo errore, che solo in parte è stato corretto, e ad equiparare per il futuro il trattamento dei titolari delle polizze vita cosiddette dormienti che non riscattano la polizza perché spesso non ne sono a conoscenza, a quello dei beneficiari dei conti correnti dormienti, in merito a prescrizione e diritto di informazione. Signora

questo documento sia in linea con molte delle tematiche difese da sempre dalla Lega Nord. Pensiamo, per esempio, all'articolo 2 che riguarda l'adeguamento della direttiva Ecofin. L'aspetto preso in esame riguarda, in primo luogo, le notifiche ai contribuenti non residenti in Italia, che si considerano validamente effettuate con la spedizione della raccomandata all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. Oltre a questo tema vediamo anche che questo articolo vuole dare un taglio netto ai cattivi amministratori. Noi della Lega Nord lo diciamo da sempre: anche nella riforma in materia di federalismo fiscale ci siamo battuti affinché chi amministra sia totalmente responsabile di qualsiasi sua azione, che nel caso sia fraudolenta deve essere assolutamente punita. Come ha già esposto il relatore senatore Casoli nella sua relazione, volevo fare notare come nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nel quale si prevedono disposizioni volte a garantire il rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di «concessioni «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali», si rilevi l'opportunità di specificare adeguatamente a quale tipologia di concessioni pubbliche si fa riferimento, tenuto conto che le disposizioni del comma 2 e dei commi successivi riguardano specificamente il settore dei giochi. Quindi, anch'io mi permetto di suggerire di delimitare la tipologia di concessione pubblica statale come relativa al settore dei giochi anche al primo periodo del comma 2. Vorrei sottolineare come in una delicatissima fase storica in cui i tassi di interesse continuavano a salire, questo Governo sia intervenuto fissando il tetto al 4 per cento per gli interessi variabili dei contratti di mutuo. Abbiamo poi istituito *social card* per gli acquisti di prima necessità, attribuita ai cittadini italiani, e il *bonus* per il pagamento dell'energia elettrica e del gas, senza tralasciare la moratoria sui mutui, essenziale strumento per garantire di superare gli effetti, purtroppo per molti, della perdita del lavoro in questo momento di crisi. Innumerevoli sono stati anche gli interventi governativi a favore delle imprese: ricordo, solo per citarne alcuni, 10 per cento dell'IRAP dall'IRE, o la concessione della rivalutazione degli immobili iscritti a bilancio a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva e così via. È importante sottolineare l'impegno del Governo anche e soprattutto sul tema del contrasto all'evasione fiscale. Con questo provvedimento, infatti, viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi appartenenti alla cosiddetta *black list,* al fine di rafforzare il contrasto ai fenomeni di evasione e di frode nel settore IVA. Tale misura è coerente con i più recenti indirizzi dell'Unione europea, volti appunto alla progressiva armonizzazione della normativa su tale imposta. Altro aspetto importante, che ha visto un nostro grande impegno come Lega Nord, è l'articolo 4, che riguarda le agevolazioni sulla ricerca nel settore tessile. In questo caso viene escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività previste alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO e cioè: ricerca e ideazione estetica; realizzazione dei prototipi; preparazione del campionario o delle collezioni; promozione del campionario; gestione del magazzino campioni. Per quanto concerne il meccansimo di applicazione, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa e opera indipendentemente dal conseguimento di reddito imponibile. Proprio con l'intento di sostenere le imprese del settore tessile e ridare un nuovo impulso alle iniziative di tutela del *made in Italy* è stato accolto alla Camera un emendamento della Lega Nord che attraverso l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze assegna alle imprese che volontariamente applicano la legge sulla commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri un contributo di cinque milioni di euro, con la finalità di sostenere il sistema di etichettatura dei prodotti. Passiamo poi all'articolo 5: qui vengono liberalizzate, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie quali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. Meno vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, agricola, per le serre mobili stagionali, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La norma fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Si prevede, poi, che al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Gli interventi, quindi, previsti dall'articolo possono essere iniziati previa semplice comunicazione anche per via telematica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori. Per concludere, credo sia necessario anche accennare ad un discorso che ritengo molto importante, quello della banda larga, dove, sempre all'articolo 5, si sono volute semplificare le procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Per tali opere, attualmente, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Il nuovo testo prevede la possibilità di ridurre comunque la profondità di scavo, a condizione che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo attività che, secondo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve essere presentata all'amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. Concludendo, l'obbligo di comunicazione può essere escluso, tramite decreto del Ministro dell'economia di natura non regolamentare, per alcuni Paesi appartenenti alla *black list* e, viceversa, può essere esteso anche a Paesi che non rientrano in tale elenco e, più in generale, anche a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti a particolare rischio di frode fiscale.

al credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione: credo che questa sia una contraddizione in termini. Permettetemi di dire che non ha

di euro al credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione. Questa è la prima assurdità: proprio una contraddizione in termini. Vengo ora invece

Mi riferisco ai 30 milioni di euro inseriti dalla Camera per ripristinare le tariffe postali agevolate per l'anno 2010, modificate con una norma che non stava né in cielo né in terra (scusate l'espressione, forse inadeguata all'Aula del Senato).

avete inserito 30 milioni di euro per la stampa *no profit*, escludendo però le riviste vendute in abbonamento da enti, sempre *no profit*, con particolare riferimento a quelle legate ad ambiti religiosi, le riviste diocesane

questa norma fa male, mette il bavaglio e toglie la possibilità di avere un confronto davvero democratico. Credo che anche voi riceviate molte riviste di quelle associazioni, preziosissime, esistenti sul nostro territorio.

era firmato dal Capogruppo della forza di maggioranza relativa nel Paese, e non era firmato dai cattocomunisti dell'opposizione, o dai radicali dell'opposizione. Ripeto: era firmato dal Presidente

il provvedimento in esame dispone importanti misure che riguardano in particolare il contrasto alle frodi fiscali finanziarie internazionali e nazionali, la razionalizzazione della riscossione, interventi agevolativi a sostegno della domanda ed il potenziamento dell'amministrazione finanziaria. Intenzione del decreto è stata, *in primis*, quella di non pregiudicare gli equilibri di bilancio e dunque di non aggravare ulteriormente il debito pubblico, evitando così di intaccare il nostro sistema finanziario nazionale, messo in sicurezza grazie alla manovra triennale del 2008. Non dimentichiamoci che la politica economica varata ha portato il nostro Paese a mantenersi in equilibrio, per quanto concerne il debito pubblico, rispetto alla Germania, e ad ottenere una posizione migliore nei confronti di altre Nazioni, compresi anche gli Stati Uniti d'America. I vari organismi internazionali (Fondo monetario internazione, Unione europea e OCSE) hanno ritenuto giusta la politica economica del Governo, nonostante la crisi globale del mercato mondiale. Il decreto in questione, nel solco di questa politica economica, si pone in una soluzione di continuità con i provvedimenti anticrisi varati dal Governo Berlusconi. In particolare, si dà continuazione a quanto disposto dal decreto-legge n. 5 del 2009, che ha introdotto misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, facendo però - in questo caso - un'operazione di rafforzamento di contrasto all'evasione fiscale, al fine di consolidare ed aumentare il gettito tributario. II decreto-legge oggi all'attenzione dell'Aula, inoltre, cerca di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Infatti, non casualmente, sono stati interessati i settori degli elettrodomestici in generale, delle cucine componibili con elettrodomestici efficienti, gli immobili con alta efficienza energetica. Dunque, ci si è rivolti a quella filiera che fa capo al bene primario degli italiani: la casa. Si sono, inoltre, tenute in considerazione le esigenze dei giovani con misure concernenti motocicli, motocicli elettrici ibridi ed Internet veloce. Tutto ciò comporta ricadute favorevoli per le aziende. In questi casi si è volutamente cercato di sostenere la domanda, dando un supporto finanziario direttamente ai consumatori ed indirettamente alle imprese. Molteplici sono state le misure di incentivazione messe a disposizione delle imprese con il provvedimento in esame. Per non dilungarmi e fare una sintesi, desidero, su questo argomento, ricordare gli interventi in favore dei distretti del settore tessile ed abbigliamento, che reputo importanti anche alla luce della politica di tutela e valorizzazione del *made in Italy*, portata avanti con forza dal nostro Governo; interventi che sono stati in seguito estesi anche al settore della fabbricazione di articoli in pelle e simili. In particolare, mi vorrei soffermare sulla situazione concernente il comparto delle calzature, settore che nella mia Regione - le Marche - riveste un'importanza economica e sociale di rilievo, poiché tantissime aziende (soprattutto piccole e medie) insistono in quel territorio ed hanno fatto conoscere a livello internazionale la creatività degli operatori e la qualità della calzatura italiana. Tale settore, in un primo momento, era stato escluso dagli incentivi previsti nel decreto in questione, per poi rientrarvi a seguito della richiesta delle categorie, richiesta accolta anche su pressione di noi parlamentari marchigiani. Mi rammarico, però, del fatto che non sia stato espressamente previsto l'inserimento di un comparto che sostanzialmente è parte integrante della filiera delle calzature e della pelletteria, ossia di quel codice 15 della tabella ATECO. In particolare, mi riferisco ai codici 22.19.01 e 22.29.01, sottovoci che fanno riferimento al settore delle suole, dei componenti e degli accessori delle calzature, che con la presentazione di un apposito emendamento ho chiesto di includere nel provvedimento in esame per non far insorgere controversie interpretative. Sono certo che che il Governo saprà venire incontro alle esigenze di questo settore, secondo quanto previsto nell'ordine del giorno presentato dal relatore insieme al sottoscritto e ad altri colleghi, dando indicazioni interpretative all'Agenzia delle entrate affinché, nello stabilire criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni, venga interpretata la norma che ha previsto la tabella 15 come rivolta all'intero comparto della calzatura, comprese - dunque - le sottovoci riferite ad accessori, suole e componenti, tutte lavorazioni indispensabili per la produzione delle scarpe. Da quanto su indicato è evidente che il Governo ha voluto dare un impulso a quelle filiere produttive già interessate dal decreto-legge n. 135 del 2009, poi convertito dalla legge n. 166 del 2009, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere con maggiore incisività il marchio del *made in Italy*. In ultima analisi il provvedimento sugli incentivi è motivato anch'esso dall'esigenza di varare misure di contrasto alla crisi prodotta da una finanza del tutto virtuale che si autodefiniva innovativa, crisi che sta interessando l'intero pianeta. Una crisi, di cui allo stato è difficile prevedere il termine, e che vede gli organismi internazionali alla ricerca spasmodica di soluzioni. In questo, la politica economica attuata dal Governo può essere d'esempio. Quella politica di rigore, responsabile, ma allo stesso tempo coraggiosa, che guarda lontano pur consapevole delle difficoltà di una ripartenza. Questo è lo spirito dell'azione del Governo Berlusconi, che è ormai presa ad esempio da altri Paesi. È palese il risultato positivo di questa politica economica, che ha saputo contrastare la crisi con provvedimenti sia pur di carattere congiunturale che non hanno mai abbandonato la logica dello sviluppo. Possiamo, dunque, affermare di aver realizzato un modello da seguire, che ha privilegiato una politica di rigore dei conti pubblici, supportato da quel grande patrimonio delle famiglie italiane che vede nel risparmio e nell'economia reale delle piccole e medie imprese due baluardi che hanno fatto grande l'Italia. Con questo decreto-legge si continua sulla strada del contenimento del debito pubblico e si pongono basi sempre più solide per accelerare la ripresa della nostra economia.

inoltre la deflazione nel contenzioso della giustizia tributaria - il che non mi sembra malvagio - e l'accorciamento dei processi tributari, senza arrivare terzo grado di giudizio;

Ho sentito ieri osservazioni molto giuste da parte dei colleghi della maggioranza, soprattutto dal senatore Conti, ed anche di alcuni senatori dell'opposizione, che mi sono sembrati sulla stessa linea, sapendo bene che

le armi che abbiamo - visto che purtroppo sono abituata a parlare di difesa - sono queste. Non so quante altre armi vi possano essere per combattere questo tipo di guerra all'economia e al nostro debito, che è uno dei più grandi del mondo.

degli enti multilaterali, che spesso si dimenticano, ricordandosi solo quelli militari; per il 2011, al rifinanziamento del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, a decorrere dall'anno 2012, alle esigenze di finanziamento Il provvedimento in esame trova quindi maggiori entrate, in questo caso, che affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e credo che chi penserà l'anno prossimo a questo Fondo

né con poco, né con troppo, semplicemente con le giuste persone, senza troppi aerei, magari con un po' più di *intelligence.* Con qualche uomo in più e con qualche uomo del SIMIC in più,

e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list,* ovvero attività lì svolte. Credo che questo sia

al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. Tutte queste *black list* e persone che escono dal nostro territorio o danno fondi all'estero e sono italiani, ritengo non debbano rientrare in Italia con passaporto italiano. Ritengo che chi desidera continuare ad essere italiano debba rientrare ad essere italiano dando se stesso, la propria vita, i propri averi, dimostrando, dall'alto al basso, quindi dal Presidente fino all'ultimo operaio, di voler fare qualcosa per il proprio Paese, e non al di fuori. Purtroppo spesso e volentieri tutti parlano, tante persone parlano una contro l'altra, e poi a lavorare sono in pochi.

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo ad affrontare la discussione di questo decreto‑legge in un momento ed in un contesto particolarmente delicato, critico e preoccupante. Il decreto reca disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali, in materia di riscossione tributaria e in materia di finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno alla domanda. Siamo ormai fuori tempo massimo per soffermarci a commentare la parte che riguarda il sostegno ai consumi e gli incentivi, interventi annunciati in pompa magna a fine 2009, rimandati o ritardati per essere approvati pochi giorni prima delle elezioni regionali, del tutto inadeguati a realizzare una seria politica economia e industriale, con poche risorse per troppi obiettivi, risorse talmente esigue da essere già, in pratica, esaurite. Un vero e proprio spot elettorale dunque che, come ogni propaganda, occulta pezzi di verità come, ad esempio (lo ha accennato la senatrice Fioroni), la sottrazione di risorse destinate al credito d'imposta per ricerca e innovazione, con ciò rovesciando le priorità di questo Paese. Ma del resto a questo ci avete abituati in questi due anni. La pervicacia con cui avete voluto evitare qualsiasi confronto e discussione di merito sui problemi reali del Paese, sui suoi ritardi strutturali, sulle politiche da mettere in campo per costruire una risposta credibile alla crisi e guidare la ripresa ha, di fatto, paralizzato l'attività di questa Aula, nonostante le nostre continue dichiarazioni di disponibilità e le nostre reiterate sollecitazioni in tal senso. E così si è consumata la più grave distorsione del ruolo stesso del Parlamento, e sotto il vestito delle tante permesse annunciate e delle molte attese indotte, il nulla, se si esclude la pericolosa assenza di una vera politica per le imprese, per il lavoro e per le famiglie, l'assenza di una politica industriale e di processi di innovazione del sistema produttivo. Ora però la maschera è caduta e in questi giorni la situazione del Paese si è presentata con il suo vero volto. Tanti richiami, ora, al rigore nei conti pubblici come priorità nell'azione di Governo. Richiami giustissimi sui quali c'è stata, c'è e ci sarà sempre da parte nostra massima condivisione. Questa è stata, peraltro, la bussola che ha contraddistinto le scelte dei Governi di centrosinistra di questi ultimi 15 anni. Ma il tema del rigore dei conti pubblici si riallaccia all'altro grande tema, quello dell'evasione ed elusione fiscale. In un Paese come il nostro, con almeno 100 miliardi di euro di evasione fiscale, con il suo carico di economia sommersa, di concorrenza sleale, di corruzione, di frode, il tema della trasparenza, delle regole, del contrasto all'illegalità diventa sempre più pregnante. Mi ricollego allora alla prima parte del decreto-legge oggi in esame, quella cioè che riguarda il contrasto alle frodi fiscali. È una piacevole sorpresa notare che il Governo ha rivisto la sua posizione, dopo aver inizialmente abolito e demonizzato tutte le misure antievasione volute dal Governo Prodi. Non possiamo far altro che apprezzare questo cambio di direzione, dopo che il primo provvedimento del ministro Tremonti nel 2008 fu proprio l'abolizione dell'invio degli elenchi clienti e fornitori, in quanto considerato vessatorio e superfluo. Nell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame almeno quella misura viene reintrodotta: un segno evidente di quanto fosse demagogica e pretestuosa la posizione di allora. Certo, ora non si capisce perché l'adempimento sia parziale e limitato a singoli settori discrezionalmente decisi dall'amministrazione per le sole transazioni con operatori economici domiciliati in Paesi della cosiddetta *black list*, quasi che vi sia una bilancia di giudizio diversa, con due pesi e due misure differenti; di questo ha però parlato in maniera approfondita il collega Barbolini. Nel provvedimento risultano esservi anche alcune misure che non vanno certo nella direzione della trasparenza e della chiarezza. Mi riferisco ai procedimenti tributari pendenti presso la Corte di cassazione, estinguibili con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia da parte del contribuente che pure risulta vincente nei primi gradi di giudizio. Mi riferisco all'esclusione degli obblighi antiriciclaggio per i gestori di alcune tipologie di giochi, tra cui Lotto, lotterie, «Gratta e vinci» e concorsi pronostici. Mi riferisco ancora al differimento del termine entro il quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avrebbe dovuto avviare la procedura per l'affidamento in concessione della rete telematica per la gestione del gioco *on line*: aspetti sui quali abbiamo chiesto chiarimenti in sede di Commissione, richiesta che ribadiamo oggi, e per i quali abbiamo presentato appositi emendamenti, sui quali però, nelle condizioni surreali del Parlamento, sappiamo rischia non esserci alcuna seria discussione. Siamo tutti consapevoli che saremo chiamati ad affrontare nel breve prove difficili per risanare la finanza pubblica e, contemporaneamente, per coniugare rigore e politiche di sviluppo. Il senatore Conti ci ha richiamato alla prossima occasione di confronto, che dovrà essere costruttivo e serio; siamo d'accordo, ma - per inciso - spiace dover dire ancora una volta che che anche in tal caso sono purtroppo i giornali e le televisioni a dare conto in questi giorni delle misure che il Governo intenderebbe assumere con la prossima manovra. Mi auguro che, effettivamente, si possa aprire quella fase che il senatore Conti richiamava. Comunque, il Gruppo del Partito Democratico farà la sua parte e formuleremo con responsabilità le nostre proposte e i nostri giudizi, ma credo che sarebbe economicamente, socialmente ed eticamente inaccettabile, iniquo ed insostenibile non mettere al primo posto il tema di una seria ed incisiva lotta all'evasione fiscale, facendo invece ricadere il costo della manovra ancora sui lavoratori, sui pensionati e sulle tante imprese oneste. Sono risposte che dovrete dare non tanto a noi, quanto ad un Paese che esige e reclama correttezza, giustizia, legalità ed equità; ad un Paese che esige e reclama una classe dirigente e politica all'altezza di questo momento.

un importante tassello di un insieme di iniziative che il Governo ha voluto promuovere a favore di tutte quelle imprese che nel corso degli ultimi mesi hanno particolarmente Ricordo che il Governo Berlusconi già nell'autunno del 2008, quando iniziarono ad acuirsi i primi segnali della crisi, intervenne con una serie di misure; innanzitutto, con la tutela dei risparmiatori e, successivamente, con un insieme di iniziative. In primo luogo, con il decreto‑legge incentivi dell'aprile 2009 che, sotto forma di sostegno alla domanda,

Il mercato dell'auto in questi ultimi mesi ha interrotto un *trend* estremamente positivo, dovuto agli incentivi, durato circa 10 mesi, e segna

La Francia invece ha una situazione migliore, in quanto il *bonus* è ancora in atto e il mercato, sia pure un po' ridimensionato, ha dato un segnale positivo dell'1,9

Il gruppo FIAT, per parlare della nostra principale azienda automobilistica, deve naturalmente fare i conti con la discesa della domanda, in relazione alla fine degli incentivi, del mercato italiano e anche di quello tedesco

con una quota di mercato a livello europeo che si attesta al 7,6 per cento, sostanzialmente in linea con i dati dei primi mesi dell'anno. Il Lingotto sottolinea come i risultati del mese alle spalle si rafforzino, con un aprile che ha aumentato le quote di mercato. Credo che dall'andamento delle vendite europee, come commenta il Centro Studi Promotor, emerga con grande chiarezza che sono gli incentivi statali a fare la differenza. In mancanza di mutamento di politica degli incentivi,

che ha portato al nostro esame il pregio e l'opportunità di destinare circa 300 milioni di euro ad una molteplicità di comparti

riguarda il fatto che le risorse previste per questo decreto non sono in grado di soddisfare interamente le istanze provenienti dai vari settori (la critica più ricorrente è quella secondo la quale le risorse sono già praticamente esaurite), non si può però mancare di osservare come nell'attuale scenario internazionale, caratterizzato da politiche economiche particolarmente restrittive ed attente al rigore nella gestione dei conti pubblici, l'intervento governativo possa risultare comunque molto apprezzato, non solo dai consumatori direttamente destinatari di incentivi sui prodotti acquistati, ma anche da tutte quelle imprese che hanno visto proprio negli ultimi mesi aumentare sensibilmente le proprie vendite in virtù dell'intervento governativo. È un elemento che voglio mettere in dovuta in dovuta evidenza e che, a differenza di quello che sostiene, come è normale che sia, l'opposizione, questo provvedimento, sia pure nella sua ristrettezza e per i motivi che più che più volte sono stati citati, ha il pregio di inserirsi nel filone di un provvedimento che avevamo già - come ho detto - approvato, che era quello sul *made in Italy*. Tutto questo nell'ottica di un'ipotesi e di una volontà di definire una politica industriale del nostro Paese che deve misurarsi con delle sfide estremamente difficili: riferisco alla crisi economica di tutto l'Occidente rispetto all'emergenza di Paesi come la Cina e l'India, e alla crisi del settore manifatturiero rispetto ad un *welfare* dell'Occidente che rimane un elemento

vanno o cominciano ad andare in quella direzione: cito per tutti l'aspetto legato alla sanità. Il nostro sistema sanitario è universalistico, è un punto di orgoglio che però comincia ad avere difficoltà nel trovare le risorse per essere finanziato: perlomeno deve necessariamente essere riorganizzato e razionalizzato per poter continuare a fornire i servizi ai nostri cittadini. Voglio ricordare, in conclusione

per garantire l'applicazione della normativa di cui al Regolamento comunitario n. 1234 del 2007, concernente i produttori vitivinicoli di alcuni prestigiosi consorzi, promotori di eccellenze, che dovrebbero essere sempre più tutelate anche nei mercati internazionali, dove la globalizzazione ha portato con sé, purtroppo, il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani che tutto il mondo ci invidia. Credo sia opportuno porre un'attenzione particolare a questo settore, che rappresenta

negativo, e lo motiverò cercando di fare qualche considerazione seppur molto rapida di politica industriale. Il provvedimento si dovrebbe inserire, almeno in parte, tra quelli di politica industriale, cioè di quella parte della politica economica che dovrebbe sostenere la competitività delle nostre imprese, la capacità delle nostre imprese di stare sul mercato e di affrontare una fase di crisi così pesante come l'attuale, che - lo voglio dire in sintesi - sta colpendo soprattutto la piccola e piccolissima dimensione d'impresa. Si parla di deficit occupazionali. Vorrei ricordare che nel 2009 (dati ISTAT) ci sono 600.000 nuovi disoccupati; di questi, 400.000 sono lavoratori autonomi: artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, liberi professionisti, per i quali non vi è alcuna forma di sostegno al reddito, nessun ammortizzatore sociale. nessuna forma, né ordinaria, né in deroga, che possa intervenire per chi è autonomo nella vita imprenditoriale o nella vita professionale. In una fase come questa sarebbero serviti provvedimenti

perché il capitale non è stato investito a fianco del lavoro e perché a bassi salari, che hanno condizionato la domanda, non è corrisposto un investimento di capitale tecnologico che aumentasse la produttività e la competitività del nostro sistema. Vi sono provvedimenti in questo disegno di legge che attengano a tale argomento? Neanche uno. Il tema della cumulazione del capitale e dell'induzione all'investimento di capitale all'interno delle imprese è ormai giudicato da tutti gli economisti e da tutti gli operatori economici un tema fondamentale di politica industriale. Vi è qualche provvedimento che induca all'investimento di capitale proprio delle persone e delle famiglie all'interno dell'impresa? Nessun provvedimento va in questa direzione. I mercati che funzionano meglio sono quelli che si liberalizzano, che aprono alla concorrenza. Vi sono provvedimenti che vanno in questa direzione? No. Devo ricordare che le tariffe dell'energia, quelle regolamentate, sono aumentate di tre punti e mezzo quelle dei mercati liberi sono aumentate di un punto e mezzo: vuol dire che la regolamentazione rappresenta un costo di sistema, che induce una scarna competitività del nostro sistema imprenditoriale. Voglio aggiungere che questi mercati non sono liberi e lo dimostra anche il Senato, quando affronta la riforma della legislazione forense, introducendo nuovi vincoli all'ingresso, l'impedimento alla costituzione di società, l'impedimento all'accesso alla professione da parte dei giovani, le tariffe minime che garantiscono lo *status quo*, la protezione dello *status quo*. Stiamo rispondendo ad una crisi globale - che viene nell'età della telematica e che si dice causata dagli squali di Wall Street Street - con misure medievali, alzando gli steccati per i garantiti e per le corporazioni, togliendo i ponti levatoi di comunicazione con i mercati e pensando di agire proteggendo un piccolo mondo antico davanti ad un mondo che è vero che propone delle sfide, ma che propone anche, se le si volessero cogliere, importanti sollecitazioni e importanti opportunità. Con questa misura non si affrontano, coerentemente come si è fatto in questi due anni, le necessità che la crisi economica ha proposto. Finiamola di raccontarci che la crisi economica è stata posta da una straordinaria crisi internazionale. La straordinaria crisi internazionale in un Paese come il nostro è ricaduta su una scarsa produttività, su una scarsa capacità competitiva del sistema, sulla sostanziale tendenza a lasciar solo il sistema produttivo rispetto a tutte le sfide cui facevo cenno prima. Perdiamo sei punti e mezzo di prodotto interno lordo negli ultimi due anni.

Era una crisi prevedibile quella internazionale? Diciamo che non lo era, anche se devo dire che il *guru* che abbiamo a fare il Ministro dell'economia avrebbe dovuto prevedere quello che è successo negli altri 15 Paesi al mondo, che nei 15 anni precedenti hanno avuto fallimenti e *default* di Stato. Diciamo che quella crisi non poteva essere prevista, perché era una crisi generata dai pigmei di Ginevra o di Zurigo, come si diceva una volta. Eppure quella crisi poteva essere affrontata in un altro modo.

È stata una contrazione dovuta alla paura, alla preoccupazione delle famiglie italiane per i propri risparmi e delle imprese per gli investimenti, a fronte di uno scenario internazionale nel quale si sentivano sole e non accompagnate dallo Stato.

bisognava evitare che si arrivasse ad una crisi della domanda da disoccupazione. L'intervento del Governo avrebbe dovuto essere forte in quel momento, non sarebbe stato uno spreco il non far collegare la paura con la disoccupazione: si trattava di sostenere la domanda e quindi il prodotto interno lordo. Adesso scopriamo che dobbiamo contenere i conti pubblici. Contenere i conti pubblici vuol dire - come avviene in ogni famiglia quando le entrate sono minori delle uscite - contenere le uscite. È doveroso, ma i conti pubblici non sono sotto controllo: la spesa intermedia della pubblica amministrazione è crescente; il saldo primario è andato fuori controllo dopo quanto era stato fatto dal Governo precedente. I conti pubblici sono fuori controllo e, contemporaneamente, non si sostiene la competitività e non si fa crescere il prodotto interno lordo. Siccome si tratta di una divisione (debito su prodotto interno lordo) il debito non diminuisce, il prodotto interno lordo cala e non si agisce né sul versante del debito, né sul versante del prodotto interno lordo. Una decisione bisognerà prenderla prima o poi,

ci si sta abituando anche nel Parlamento all'idea che una crisi economica, che sta diventando anche una crisi sociale, possa sopportare contemporaneamente una crisi istituzionale. che davanti ai mercati internazionali la credibilità di un Paese è data dalla credibilità delle sue imprese e dalle regole che questo Paese dà per far rispettare l'economia; è data dalla libertà e dal trasparente funzionamento dei mercati (e non possiamo dire che da noi le cose vadano così), ma anche dalla credibilità delle sue istituzioni. Innestare un attacco alle istituzioni e continuare a favorirlo mediaticamente nel momento in cui c'è una grave crisi sociale e anche una grave crisi economica

Qui ci sono politiche economiche sbagliate: una maggiore democrazia e un maggiore confronto consentirebbe di correggerne gli effetti e i risultati.

fondamentale che il sistema, il Palazzo non dia un'immagine di ulteriori complicazioni e crisi. Tant'è che in uno dei recenti bollettini dell'agenzia di *rating* Moody's si diceva: per l'Italia tutto bene, addirittura prospettive di aumento di *rating*, però c'è il rischio istituzionale, c'è il rischio politico. Sarebbe veramente il colmo che, con tutti i problemi che abbiamo, innescassimo anche questo. da parte di tutti, in un periodo così complicato, un po' di tranquillità e pacatezza e cercare insieme di recuperare questi 25 miliardi di euro che abbiamo bisogno di trovare in fretta.

Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo ridurre i costi; e poi, se non ce la facciamo, mobilità, cassa integrazione, licenziamento, prima di arrivare al fallimento. Quindi, la via è obbligata; e allora ragioniamo insieme su dove trovare questi 25

per arrivare a 25.000 ne servirebbero di Senati della Repubblica! Quindi, non è questa, chiaramente, la soluzione, ma è giusto dare un esempio. È giusto che si dia l'esempio anche in tutti quei settori della pubblica amministrazione dove si registrano retribuzioni non legate ad una vera produttività. Al riguardo, leggendo i giornali, non esiste neanche una stima di quanti siano i dipendenti pubblici con

sostanza è che, come in un'azienda privata quando il fatturato cala prima di arrivare al fallimento si debbono ridurre i costi, così anche l'azienda Italia, prima di arrivare al fallimento, deve ridurre i costi, e uno di questi è il personale. Sul lato pensioni abbiamo già dato ampiamente; l'altra voce forte di spesa di questo Stato è la voce sanità, e è la voce sanità, e sappiamo benissimo che ci sono enormi margini di miglioramento: lo scorso anno le Regioni che hanno sforato lo hanno fatto per 3 miliardi e mezzo.

prima, di fare meglio, e quindi di farlo ancora più forte questo federalismo fiscale, perché è nell'interesse di tutto il sistema; altrimenti, lo dico semplicemente, si va a ramengo. Venendo al provvedimento, mi limito ad illustrare

su una questione molto semplice, che è un esempio di quello che dovremmo fare strutturalmente: visto che non ci sono risorse, perlomeno non facciamo perdere tempo e quattrini alle imprese.

legislativa di cui discutiamo oggi e offrire una visione comparata dell'immagine dell'Italia. Io, insieme al collega Giordano, rappresento gli italiani che vivono all'estero e ci tengo, in questa occasione, a segnalare che

Ciò è certamente merito della stabilità di governo realizzata dall'Esecutivo Berlusconi nella penultima legislatura e dell'azione di governo portata avanti in questo periodo anche attraverso interventi di questo tipo.

ascrivibili all'azione di questo Governo, hanno portato l'Italia a confermare la sua posizione non solo all'interno del G8 e dei Paesi più competitivi, ma anche all'interno dell'Europa, con il terzo PIL europeo. Abbiamo scoperto con piacere in seguito alla crisi finanziaria mondiale, attraverso i disastri causati dalla finanziarizzazione dell'economia,

che, ad esempio, in tema di bilanci pubblici, da quando vengono opportunamente presi in considerazione il settore del settore del debito pubblico e quello del debito privato, la posizione italiana comparata all'interno dell'Unione europea è fortemente migliorata. Questo è un altro merito ascrivibile al Governo Berlusconi e all'azione di governo che viene portata avanti anche attraverso

pubblici e privati relativamente più in ordine. Questo è il risultato di un'azione di governo positiva di cui ci viene dato atto anche a livello europeo, in quelle comunità che noi rappresentiamo, e di cui gli italiani all'estero residenti in Europa e non solo sono particolarmente orgogliosi. Faccio un'ultima considerazione. È di questi giorni il dato che segnala dell'*export* italiano, in particolare nei quattro settori dove le nostre piccole e medie imprese sono eccellenti e ottengono risultati che fanno onore alla nostra economia, cioè nei settori

Plaudiamo all'azione del Governo e ad iniziative di politica economica di questo genere, proprio in considerazione del fatto che ci garantiscono uno *status*, posizioni migliori

avendo un tempo limitato per essere convertiti, vanno ad una delle due Camere dove possono subire modifiche, ma in genere in seconda lettura presso l'altra Camera arrivano blindati per esigenze di tempo. In verità, nei decenni passati, nella cosiddetta Prima Repubblica, ciò poteva anche non accadere, ossia il decreto poteva subire anche in seconda Camera una modifica, perché se poi decadeva vi era l'abitudine di reiterarlo. Oggi, che viviamo in epoca diversa, nella quale ciò non sarebbe consentito dal Capo dello Stato, esiste la necessità di svolgere un dibattito, complessivamente inutile,

Ma perché andare un po' fuori le righe e fuori argomento? Perché il mondo delle imprese italiane avrebbe bisogno di essere incentivato, incentivato, soprattutto in quei tanti settori merceologici che non sono stati mai interessati da incentivi. Questi hanno tradizionalmente riguardato il settore dell'automobile, quello degli elettrodomestici, dell'energia e pochi altri ancora. Tutto il mondo produttivo italiano, che peraltro - lo ricordo - è fatto da micro-piccole piuttosto che da medio-grandi imprese, avrebbe bisogno di una attenzione particolare,

giornata di martedì prossimo. Al contrario, abbiamo un argomento all'attenzione molto più serio, a cui pure qualche collega che mi ha preceduto ha fatto cenno, ossia la prossima manovra finanziaria.

la casta della politica, che al momento è all'attenzione anche del ministro Tremonti per il noto aperitivo in cui ieri ci ha in qualche modo individuato. Sono d'accordo su tutti i provvedimenti che saranno presi per abbattere i costi della politica, sia in termini di indennità che di riduzione dei componenti dei tanti e troppi

che - ricordo - è anch'esso una casta. Ecco allora il mio andare fuori le righe. Parliamo dell'informazione che percepisce contributi per l'editoria e per le Parliamo di questo mondo dell'informazione di cui, caro Sottosegretario, ho cognizione diretta del lavoro nero che si svolge in tutte le redazioni regionali e locali anche dei massimi quotidiani dell'informazione. C'è tanto lavoro nero e precariato. Allora ecco, a me dà fastidio che chi parla in termini moralistici e non riesce ad andare oltre, ai contenuti, poi ci fa la morale

ve ne sono tante altre in Italia. Ho appreso con piacere l'intenzione del ministro Tremonti di rivolgere un'attenzione particolare al settore dell'invalidità civile.

Tremonti ha detto di volerci mettere mano, ma vorrei che il Sottosegretario, anziché essere disturbato dal relatore Casoli, mi prestasse attenzione e suggerisse, ad esempio, al ministro Sacconi di compiere

e a qualsiasi convegno abbia partecipato - e l'Italia è ammalata di «convegnite» - ho sempre pagato da me il mio conto di albergo. Sono una perla rara:

mentre leggo di queste presunte manovre di 25-27 miliardi di euro che il Governo si accinge a varare,

in parte viene dall'estero, in parte vi sono però anche gravissime responsabilità di coloro che, per due anni, hanno additato come catastrofista chi non voleva chiudere gli occhi di fronte ad un Paese che non era quello raccontato dai telegiornali e dai giornali di regime. Era un Paese che soffriva la disoccupazione, la distruzione dei posti di lavoro, il Paese di quei precari che hanno due lauree e devono sputare sangue per farsi rinnovare il contratto trimestrale. Ma che Paese ci avete raccontato in questi due anni?

Il Paese di Bengodi, dove i furbi l'hanno fatta franca, dove c'è stato il terzo scudo fiscale, dove c'è una corruzione dilagante. E oggi ci venite a dire che l'emergenza di questo Paese sono le intercettazioni telefoniche: la vostra ossessione, per togliere ai magistrati e a chi indaga uno strumento importante! Non commento quello che ieri ha affermato un sottosegretario di questo Governo, la signora Santanché, che ha detto che bisogna rispettare la *privacy* dei mafiosi. Non lo commenterò. Però ci avete raccontato un Paese che non c'era,

riuscendo ad ottenere alcune correzioni, hanno votato a favore. Non siamo quindi solo quelli del no: però non ci potete prendere in giro e non potete prendere in giro il Paese. Mi fa piacere che anche il collega Paravia

dobbiamo rilevare che esiste uno sfruttamento, una condizione davvero odiosa e presente in tantissime categorie, soprattutto nel Mezzogiorno, e che gli ammortizzatori sociali, quelli veri,

per garantire a questo Paese la competitività, voi le state smantellando giorno dopo giorno. Già ho detto dell'azione di classe svuotata, della *farce action* del ministro Brunetta. Secondo i dati

con una spocchia che non finiva più, affermando che loro sono al di sopra della legge perché i Governi democratici hanno delegato a questi oligarchi

non estorcano altro dagli Stati. Estorsione con il concorso del controllore in Italia, di quella Banca d'Italia che quando fu fatta la legge n. 108 del 1996 - vi ricordate il treno contro l'usura, gli imprenditori strozzati? Una volta c'era la condizione di bisogno, e poi il tasso soglia - disse che la commissione di massimo scoperto non doveva rientrare nei calcoli. Per fortuna, ci sono giudici a Berlino e c'è una sentenza penale della Corte di cassazione che afferma che la Banca d'Italia non può

affermando che per far ripartire questo Paese bisogna davvero tagliare gli sprechi. Lo dice anche il presidente Baldassarri: 38 miliardi di euro a fondo perduto, che non si sa che fine fanno.

quindi, la Protezione civile non doveva rispettare quelle norme su cui noi abbiamo fatto tante battaglie perché la trasparenza è amica della legalità e, invece, l'oscurità è amica dell'imbroglio. Noi siamo molto severi; non ho parlato di questo decreto blindato, dell'estorsione ai poveri vecchi, agli assicurati che avevano le polizze dormienti; non ho parlato dei 200 milioni di euro alla Mondadori e di tante altre questioni, perché questo è appunto un decreto blindato, scade. E poi si dice che il Parlamento non lavora: ma se non ci si dà la possibilità di lavorare? Chi vuole lavorare in Parlamento - uno come me lo sa - può lavorare. Noi dell'Italia dei Valori esprimiamo pertanto un giudizio davvero molto critico e ci auguriamo che il Governo operi un ravvedimento operoso e, prima di mettere le mani nelle tasche della povera gente, si rivolga almeno ai banchieri che hanno prodotto la crisi, che si sono aumentati gli stipendi, che non danno un euro alle imprese (e non sapete quante

e prendendo i soldi da questi signori banchieri, che finalmente devono pagare il conto anche loro, e non solo la povera gente e i lavoratori!

che gli avesse permesso di essere cambiato. Purtroppo, non è stato blindato soltanto al Senato, come l'onorevole Sottosegretario sa,

alla blindatura di questo provvedimento, che non ha avuto la possibilità di essere cambiato né in un ramo del Parlamento, né nell'altro. Signor

ritardo con il quale è stato adottato rispetto alle promesse e alle dichiarazioni stampa che ne avevano anticipato una parte dei contenuti, ma soprattutto per la grave inadeguatezza della modalità e della quantità di erogazioni di risorse rispetto ad un modello di incentivi che si è dimostrato poter essere un buon modello e che in pochi giorni, tra l'altro, ha già esaurito le sue risorse. Il quadro generale di finanza pubblica è sicuramente molto preoccupante: un avanzo primario ormai azzerato, un preoccupante incedere della spesa corrente, che è cresciuta di 12 miliardi nel 2009, e il *deficit* che è aumentato di 35 miliardi. La spina dorsale dell'economia italiana, ovvero la piccola e media impresa (noi contiamo 4,5 milioni di aziende e 4,5 milioni di imprenditori che tutte le mattine sono pressati da gravosi, grossi sacrifici, e aprono tuttavia le loro attività), quest'anno

importanti del nostro Paese, in crisi di ordini, in forte deficit, con difficoltà di esportazioni e, soprattutto con l'approssimarsi della presentazione dei bilanci del 2009, con una preoccupante

Sul fronte fiscale, finalmente si reintroducono strumenti contro l'evasione, sospinti anche dall'opinione pubblica, a causa anche degli eventi di recente attualità. sull'evasione si deve e si può fare di più. Oggi il Governo si è reso conto che l'evasione non è soltanto una macchia molto ampia

siano portate avanti dal Ministro e che alla fine non siano sempre i soliti conosciuti a pagare un momento di crisi. Ma la parte più deludente di questo decreto-legge è sicuramente quella legata all'assenza di una politica per le imprese. Le norme varate non incidono in modo tangibile e con effetti benefici sulla piccola e media impresa di cui tutti siamo bravi a dire che è il tessuto è il tessuto importante, la base vera e reale dell'economia del Paese. Così è successo per la proroga del modello unico di dichiarazione al 30 giugno, per la redistribuzione delle quote di emissione di anidride carbonica per i nuovi e per la proroga delle concessioni idroelettriche. Sono temi fondamentali per la competitività delle imprese che dovranno accollarsi altri costi, oltre a scontare un'incertezza delle norme. Basti pensare che l'assenza di regole certe sul modello unico di dichiarazione metterà circa 600.000 aziende che attendevano la proroga del vecchio modello di dichiarazione in una situazione di illegalità già dal mese di maggio. Lo stesso dicasi per le quote di emissione che, anche se riguardano una platea di soggetti più limitata, avranno degli effetti negativi pesanti in quanto quelle disponibili non sono sufficienti. Insomma, in questo decreto, di incentivo è rimasto solo la parola, perché definire un provvedimento in questa maniera e parlare di una somma totale per risollevare le sorti delle imprese del nostro Paese di circa 25-30 milioni di euro è una contraddizione in termini. In un momento come questo tale quota di incentivi sarebbe bastata per un unico settore che oggi è in crisi, qualsiasi settore: allora, a questo punto, ci sarebbe stata oggettivamente una risposta da parte del Governo. Abbiamo sperato che alcune proposte emendative di buon senso venissero accolte, ma non solo qui al Senato: parlo anche della Camera perché queste proposte di buon senso sono state respinte alla Camera sia in in Aula. Non vi è stato alcun atteggiamento di disponibilità nei confronti dei pochi, pochissimi emendamenti che abbiamo presentato, volendo anche con questo togliere il Governo dall'imbarazzo di apporre l'ennesima questione di fiducia su un provvedimento che poteva avere sicuramente una diversa portata. E noi speriamo che il Governo non ponga almeno la fiducia. Gli emendamenti presentati e non accolti riguardano per esempio la rottamazione delle caldaie per il riscaldamento: ci sembrava una cosa buona e giusta per le famiglie e per le aziende che investono in questo tipo di settore; o la rottamazione delle macchine agricole, anche in virtù di una sana politica per l'ambiente (si parla tanto di riprendere l'agricoltura come forza trainante della nostra economia, però ascoltiamo solo delle parole). Non è stato approvato un emendamento che parla della dilatazione dei pagamenti per le imprese nei confronti del fisco, quando c'è una difficoltà seria ad onorare questo tipo di imposta, per un massimo di dodici mesi quando l'importo è superiore ai 250.000 euro. Anche questa ci sembrava una proposta di buon senso: abbiamo assistito a sanatorie con rientri di capitali dall'estero ad un tasso veramente veramente banale; prevedere una dilatazione per un anno per le imprese in difficoltà nei confronti del fisco con una rateizzazione forse sarebbe stato un segnale di vera attenzione a quelle aziende che appunto si trovano in difficoltà. Non è stata data alcuna attenzione all'imprenditoria femminile. Non vi è traccia nemmeno di qualcosa che a noi sta tanto a cuore: sto parlando delle piccole imprese familiari, perché anche lì si poteva dare un segno chiaro e forte di attenzione. Tutti parliamo di famiglia, di imprese familiari salvo poi dimenticarle puntualmente quando vi è la possibilità di incidere con provvedimenti come questo. Signora Presidente, concludo esprimendo ovviamente un parere critico su questo provvedimento, che poteva essere una grande occasione che ancora una volta il Governo ha perso.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Giorgetti, abbiamo sentito la sinistra, l'opposizione esprimere totale ed ampia contrarietà sui contenuti di questo provvedimento. Quindi, è giusto forse anche ricordare quali sono i contenuti di questo provvedimento. Sono il contrasto delle frodi fiscali; incentivi come misure anticicliche per sostenere le imprese e mantenere il consumo delle famiglie e dei giovani e quindi non ledere i bisogni di queste categorie.; sono incentivi come misure strutturali proiettate al futuro per le imprese, per abbattere i consumi energetici, ad esempio, e quindi non solo per ridurre i costi diretti, ma anche indiretti, se si pensa agli effetti positivi ambientali che hanno questi provvedimenti; sono semplificazioni di procedimenti amministrativi, quindi con minori costi e con maggiore chiarezza e trasparenza verso i cittadini e le imprese; sono la liberalizzazione delle attività edilizie per particolari e semplici opere che hanno effetti positivi per le imprese fruitrici e le imprese esecutrici. Il fatto importante in questo provvedimento è poi che questi incentivi, questi strumenti sono finanziati proprio con il contrasto alle frodi fiscali e quindi in modo assolutamente virtuoso e positivo.

non la maggioranza e non la Lega Nord. Certo, si può fare di più e meglio. Questo ovviamente è uno stimolo che deve spingere sempre tutti gli amministratori e che ci spinge e ci sostiene in ogni nostro intervento. Ma questo sarà possibile, come ha ricordato il senatore Massimo Garavaglia, con il federalismo fiscale. Ormai, infatti, questo Stato è arrivato al fondo delle sue capacità di dare una risposta forte e strutturale. quindi, voglio invitare tutte le forze politiche a sostenere le riforme per le quali la Lega Nord da sempre combatte, su richiesta e su spinta dei cittadini. Desidero intervenire, inoltre, sul tema delle imprese familiari che, insieme alle piccole e medie imprese, sono la spina dorsale sana ed economicamente virtuosa del nostro Paese.

imprese di famiglia alla seconda generazione le prime tre Regioni sono, in quest'ordine, il Trentino-Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Piemonte tre Regioni d'Italia sono il Molise, l'Abruzzo e la Basilicata. Se andiamo, poi, alle imprese di famiglia di terza generazione, vediamo come prime tre Regioni, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte e come ultime tre la Calabria, l'Abruzzo e il Molise. Passiamo, quindi, alla statistica che ci mostra i dati sulle imprese di famiglia di quarta generazione:

ed esportata in tutto il resto del Paese, se riteniamo veramente, come molti dicono, che sulle piccole e medie imprese e sulle imprese familiari vanno previsti i giusti investimenti e sostegni, pur, ovviamente, in un mercato che riconosciamo essere globale e che deve vedere quindi anche una concertazione e una capacità di unione delle imprese, che può essere attuata con altri strumenti, quali i lavori dei distretti o dei consorzi. Sulla necessità, quindi, di tener conto di queste diversità del nostro sistema Paese e sulla necessità di far sì che vi siano questi sviluppi sui vari territori ho presentato anche un disegno di legge alle zone franche, le mie zone di montagna, per un rilancio economico e per evitare che vi sia lo spopolamento, che comporta costi per il sistema generale. È importante mantenere le persone a vivere e operare dove nascono, dal momento che conoscono la cultura, la tradizione e i luoghi. Potrebbe anche essere utile ragionare su un provvedimento finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma ad esempio di credito d'imposta, il rientro in Italia di cittadini comunitari.

affrontiamo questo dibattito con lo sguardo rivolto agli impegni che ci attendono: il decreto sulla Grecia la settimana prossima e, soprattutto, la pesante manovra correttiva dei conti. Per affrontare con responsabilità gli impegni futuri ci serve però un giudizio chiaro sul passato: lo dico al senatore Massimo Garavaglia, perché condivido la sua analisi, di guardare a quelle scadenze. Per noi il passato è fatto di gravi inadempienze e imprudenze da parte del Governo. Lo dimostra questo decreto: è stato presentato il 25 marzo, non qualche mese fa, quando vi erano tutti gli elementi per valutare comunque le pesanti conseguenze che la crisi lasciava sulla finanza pubblica, sulla capacità competitiva delle imprese e su un'impennata purtroppo non transitoria della disoccupazione; vi erano tutti gli elementi per valutare i rischi di un ulteriore peggioramento. Eppure la risposta del Governo è stata questo decreto, dai contenuti esili e inconsistenti, e la negazione assoluta fino a qualche giorno fa di ogni necessità di manovra correttiva. Il senatore Garavaglia afferma che quando le imprese sono in crisi si deve operare sulla struttura dei costi e sui tagli (questo senz'altro, qualche volta si cambia anche l'amministratore delegato, se non ha raggiunto il *target*, o si cercano nuovi prodottti*)*: perché non lo avete fatto finora? Il 6 maggio il ministro Tremonti ha presentato la prima tabellina, a pagina 1, ci conferma che il debito pubblico passa in un anno, tra il 2008 e il 2009, dal 106,1 per del PIL: sono 9,7 punti di PIL. Certo, l'abbassamento del PIL influisce sull'innalzamento del rapporto a parità di spesa, ma il problema è che le spese sono enormemente aumentate: altro che taglio delle spese! In un solo anno avete speso 6,9 miliardi di euro in più solo per i consumi intermedi e le altre spese correnti, quello che serve a far funzionare la macchina dello Stato oltre agli stipendi: un'enormità, che dimostra il fallimento che non potevate ignorare. Non è una novità della Grecia: non lo potevate ignorare nel controllo della spesa corrente. E mentre i rubinetti della spesa centrale erano spalancati avete riversato sulla spesa locale gli oneri del contenimento. Altro che federalismo! Avete fatto finta di niente perché non si doveva turbare la rappresentazione di un Paese senza problemi in cui la crisi era superata. L'altro L'altro ieri il ministro Bossi nel Veneto ha detto che non possiamo perdere l'euro, è l'unica moneta di scambio che abbiamo; con cosa pagheremmo dopo? Giusto. Se fosse stato interamente onesto avrebbe dovuto aggiungere: «Ringrazio perciò Prodi e Ciampi, che prima di noi hanno capito come stavano le cose e ci hanno salvato dotandoci, contro il nostro parere» - della Lega e dell'opposizione di allora - «della protezione dell'euro». Ora la propaganda è finita. Non si possono sostituire alle misure necessarie le brillanti chiacchierate del Ministro dell'economia, com'è stato fatto fino all'autunno scorso (poi il Ministro ha capito che le chiacchiere non bastavano più). Ve lo abbiamo detto fin dall'inizio della legislatura, non ci avete ascoltato e oggi paghiamo tutti il conto di questi ritardi. Noi siamo pronti, signor Sottosegretario, nell'interesse del Paese a dare il nostro contributo, ma non pensate di cavarvela un'altra volta con provvedimenti *una tantum* tosando i soliti noti. Se ne esce in un modo solo; con un coraggioso piano di modernizzazione del Paese attorno a tre parole: equità, efficienza della spesa e, perciò, crescita. Solo così avrete e avremo tutti l'autorità necessaria per chiedere sacrifici, perché lì si chiederanno in modo equo e perché in modo equo saranno distribuiti i frutti del risanamento.

di questi cespiti all'imposta sui redditi è passato dal 52 al 70 per cento: pensiamo che siano ancora quelli che devono fare i sacrifici? Ricordo che in questa grossa perturbazione finanziaria ci sono molti che ci perdono

Sul merito del decreto, il nostro giudizio è negativo ed è stato già illustrato dai colleghi del Gruppo; faccio solo due esempi. Sul fisco: si vuole combattere l'evasione fiscale e in modo particolare l'uso dei paradisi fiscali. Bene, siamo d'accordo, eravamo contrari anche per questo allo scudo fiscale. Però lo fate con armi spuntate: viene introdotto l'obbligo di comunicare l'elenco clienti e fornitori per le transazioni con operatori residenti in Paesi della *black list*,

Ma perché non volete riconoscere semplicemente l'errore? Avete sbagliato a togliere l'elenco clienti e fornitori in un Paese ad altissima evasione IVA: riconoscete questo errore e correggetelo. È stato facile raccogliere il consenso, ma ora tutti pagano il prezzo. Se ho ancora un minuto, signora Presidente, uno solo, vorrei dire qualcosa sugli incentivi. Si tolgono 150 milioni di euro già stanziati a favore delle imprese per fare ricerca e per il fondo sulla finanza d'impresa: li prendete, li togliete alle imprese e li mettete in una sorta di lotteria che riguarda

è stato più il tempo in cui si è parlato sui giornali di queste promesse che i giorni in cui è stato in vigore il provvedimento. È questa la politica industriale di un Paese come il nostro? Un po' di spot elettorali! È uno scandalo, colleghi, che in un momento di gravissima crisi economica il Governo non abbia ancora utilizzato la delega - ce l'avete che scade tra due mesi per il riordino del sistema degli incentivi alle imprese che, quello sì, avrebbe potuto portare maggiore efficienza nella spesa e maggiore chiarezza. Non si può veramente ingannare ulteriormente l'opinione pubblica: è ora che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento per un discorso di verità di fronte al Paese. finestra"). Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giulio Adamoli» di Besozzo, in provincia di Varese, ai quali diamo il benvenuto.

il senatore Giaretta è riuscito a rispondersi da solo nel suo intervento a proposito vuoi dell'elenco clienti e fornitori vuoi di una politica industriale che invece il nostro Governo, il Governo che questa maggioranza sostiene, sta cercando di svolgere nel migliore dei modi proprio all'interno di quella delega che egli ha citato. Una delega

che deriva da un proficuo lavoro svolto nelle Commissioni del Senato e che i relatori hanno potuto rappresentare oggi molto bene, spesso con l'apporto responsabile di proposte provenienti anche dalle opposizioni, modifiche che hanno potuto integrare e arricchire il testo originariamente presentato dal Governo con nuove e rilevanti misure, che però non hanno alterato l'impianto originale che voleva interventi in quattro grandi filoni: contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali; potenziamento dell'amministrazione finanziaria; razionalizzazione della riscossione; interventi agevolativi a sostegno della domanda. Un impianto che, come hanno già ricordato molto bene i precedenti interventi, come quello del senatore Garavaglia, si pone su una linea di continuità con altri precedenti provvedimenti varati per fronteggiare questa crisi e le sue modalità. Una continuità certamente di carattere finanziario. Anche questo provvedimento, infatti, si situa «al di qua» della linea di bilancio, non fa scatti in avanti. Continua a garantire il mantenimento degli equilibri dei conti pubblici, quella scelta di rigore intrapresa fin dall'inizio della crisi e che sta premiando il nostro Paese; quella che veniva considerata pavida e insufficiente, anche un po' provinciale, molto semplice, rispetto al *glamour* dei roboanti piani di sostegno decisi da altri Paesi. È stata una scelta che però si è rivelata particolarmente oculata. Una continuità certamente delle iniziative, oltre che del profilo finanziario, volte a sostenere la ripresa economica di cui necessita il Paese, in questo momento. Quindi, giusto - così mi sembra si possa sintetizzare il giudizio che le opposizioni hanno dato nel corso dell'esame in Commissione Commissione - proseguire sulla linea di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali, e puntare a un serio potenziamento dell'Amministrazione finanziaria. Così come è giusta la decisione di prevedere incentivi per determinati settori tradizionalmente esclusi da misure incentivanti e specifiche, come ha ricordato il sottosegretario Giorgetti nella discussione in Commissione e come ha ricordato il relatore Casoli stamattina - e per quelli che potrebbero maggiormente risentire della recessione internazionale, perché esposti più da vicino alle tensioni sull'*export* della nostra economia.

misure che, insieme a quelle di sostegno ai redditi, costituiscono un *mix* adeguato al momento di crisi economico-sociale nazionale e internazionale. Coloro che si appoggiano ai giudizi esteri spesso per legittimare i propri, dovrebbero almeno prendere atto - per onestà intellettuale di quanto espresso al riguardo non dai soliti "autorevoli" commentatori o giornali, ma dagli organismi economici internazionali. Quelle misure hanno impedito al nostro Paese di intraprendere quella deriva, soprattutto sociale, prima che finanziaria, come è avvenuto per la Grecia e che potrebbe avvenire per altri Paesi europei in seguito al "contagio". Ed è proprio dal punto di vista sociale che bisognerà verificare la tenuta del piano di aiuti recentemente varato per Atene. Un piano necessario, al quale l'Italia partecipa con 1 punto di PIL, per circa 15 miliardi in tre anni. Un intervento che non può costituire un precedente "assistenzialistico" e che rappresenta anche un monito: le imprudenze hanno un costo altissimo, che pagano principalmente i più deboli. Tuttavia, signora Presidente, vorrei evitare di fornire un contributo, anche piccolo, alla inutile, quanto noiosa, polemica per cui con il provvedimento oggi all'esame il Governo oggi all'esame il Governo ha fatto troppo poco e poteva fare di più. Mi sembra più interessante, invece, sottolineare come questo provvedimento contenga iniziative, sia originarie sia apportate dal lavoro parlamentare, che per certi versi rivestono un carattere di novità. Iniziative di cui non si può giudicare il solo volano economico che rappresentano: non è solo l'impatto finanziario a fare la bontà di un provvedimento. sta nella capacità di produrre effetti benefici in campi che apparentemente sono diversi da quello proprio del decreto-legge e che si rifanno all'esigenza di efficienza e di semplificazione, ma soprattutto di modernizzazione dell'apparato. Le misure di rafforzamento dell'Amministrazione finanziaria consentiranno un più deciso contrasto all'evasione fiscale (per memoria: nel 2009 l'attività antievasione ha recuperato 9,1 miliardi, cento rispetto al 2008) poiché incidono sul riassetto complessivo di quell'Amministrazione. Come non vedere, in tal senso, il circolo virtuoso che si innesta tra il potenziamento "conoscitivo" e quello "organizzativo", con la norma che consente la massima flessibilità e mobilità delle risorse umane e il rafforzamento di quella dei Monopoli? E le misure volte a una complessiva riduzione del contenzioso tributario? Senatrice Fontana, più che risponderle sull'elenco clienti-fornitori, preferisco rispondere a questo. Fuori da falsi moralismi, appare intollerabile che siano ancora in essere contenziosi iniziati nei primi anni (ormai, quindi, nel secolo scorso) tra lo Stato e coloro che hanno esercitato servizi di riscossione, oppure che esistano ancora (davanti alla commissione tributaria centrale o alla Cassazione) procedimenti ultradecennali che sono riferiti ad imposte e fattispecie addirittura non più esistenti. In situazioni come queste, è ancora possibile parlare di giustizia? Quanto pesa tutto ciò nel cambiamento degli apparati che devono fornire forse il bene pubblico più prezioso, quale è quello della giustizia? Per non parlare della disposizione che consente di non presentare la DIA (sempre che non si metta a repentaglio la stabilità degli immobili), facilitando le ristrutturazioni edilizie, oppure di quella per cui gli amministratori delle società ammesse alle procedure per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza non possono esercitare per dieci anni le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione.

sull'efficacia e l'efficienza della macchina pubblica, sulla semplificazione e sul processo di liberalizzazione. Ritorni che, in ultima analisi, costituiscono l'obiettivo strategico dell'azione di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene e - perché no?

parola in replica anche a nome del senatore Conti, che mi dà questa delega. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi

all'innovazione e al risveglio del mercato, ma ciò non è possibile perché le risorse sono chiaramente limitate. Ritengo, però, che le scelte operate dal Governo anche nell'ambito delle polizze dormienti e delle innovazioni siano coerenti con lo stato attuale delle nostre finanze.

una soluzione di compromesso. Ma è indubbio che anche in questo caso ci troviamo di fronte a un problema di mercato. Le Poste hanno i loro costi e non possiamo assolutamente continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. A volte - questa è

vada nella direzione che il Governo e lo Stato devono seguire per affrontare i difficili momenti del futuro. Il senatore Piscitelli ha ricordato un emendamento che ha lo scopo di allargare una categoria di beni

con qualità, tirando fuori degli argomenti che sicuramente possono servire come traccia e oggi il Sottosegretario ne ha dato dimostrazione mantenendo sempre alta l'attenzione. Sicuramente potranno servire per aiutare

che vuole ridisegnare la politica industriale italiana, non ha queste pretese. Si tratta di un decreto di sostegno e di incentivazione al consumo. Il Governo sta pensando in maniera più profonda al ridisegno della politica industriale italiana. Non penso

ed incentivi. Dobbiamo tornare ad avere una politica industriale italiana - su questo si sta lavorando - che permetta al sistema industriale italiano di ritornare ad essere leader nella innovazione e nella creazione di prodotti che siano accettati

esempio di fiore all'occhiello di una partecipazione statale che ritengo abbia dimostrato, unita ad una politica internazionale industriale, di portare in Italia tante competenze e anche tante opportunità. Noi dobbiamo seguire quella traccia.

alla crisi reale. Senatore Lannutti, la ringrazio per la stima, che è reciproca: la crisi reale c'è fin dall'inizio. Con questo non dico che il Governo l'ha nascosta, ci mancherebbe altro. Secondo me, però, il Governo ha fatto in maniera molto cosciente il suo ruolo. La Nazione deve avere fiducia

negli ultimi mesi, in maniera forse un po' sconsiderata, derise e messe alla berlina su fatti che poi si sono rivelati inesistenti. Ed è questa la ragione per cui cui non pensiamo che la normativa che stiamo discutendo sulle intercettazioni sia la panacea di tutti i mali; ma riteniamo che evitare che false informazioni vengano pubblicate

Si è parlato della necessità di avere coraggio verso quelle istituzioni bancarie, quelle grandi aziende o quei grandi monopoli

sono ormai due legislature che sono in Senato e ricordo perfettamente le lenzuolate di Bersani che parlava di liberalizzazioni; ma poi, quando si andavano a toccare i risultati, erano veramente risibili. Quelli sì che erano risibili. Nei prossimi giorni in 10ª Commissione ci

e l'evocazione della necessità di un'assunzione di responsabilità collettiva sui problemi e sulle misure che verranno che dimostra, per comparazione, l'esiguità di quello di

in campo su tematiche di sostegno all'economia, che non effettivamente interventi che possano avere l'ambizione di incidere in termini strutturali e di efficacia sull'andamento dell'economia reale, sull'occupazione e quant'altro. Ritorno ai punti che andrebbero, secondo me, incorniciati per una riflessione che che non pretendo si faccia in quest'Aula, ma spero si faccia in qualche riunione più ristretta e riservata: le riflessioni che il presidente Baldassarri ha condotto sulla inconsistenza di una politica economica e industriale appoggiata su questi provvedimenti.

su accertamenti ed introiti e non sono una fotografia dell'andamento reale: invito tutti a osservare come cala l'IVA e come cala molto più di quanto non calino i consumi per avere una spia del fatto che forse le cose richiederebbero di essere approcciate con maggiore determinazione, serietà e responsabilità. Da questo punto di vista, con una mano si cerca di prendere con l'altra si continuano a lasciare scorrere proventi che potrebbero essere incamerati e introitati. Non mi ha convinto la risposta della senatrice Bonfrisco sul tema del contenzioso tributario;

però il federalismo fiscale mi sembra che in questa fase sia evocato come un mantra, sembra quasi la coperta di Linus: di fronte ad un Paese che ha tante difficoltà, conosce i problemi e rischia la stasi e la stagnazione che conosciamo, con le criticità che sono all'ordine del giorno, ogni volta si evoca il federalismo fiscale. Ebbene, facciamolo! Cominciamo, per esempio, a mettere nero su bianco gli elenchi degli immobili e dei terreni che devono essere trasferiti: non la generica individuazione del concetto, ma gli elenchi, perché da essi si capisce se

discuteremo, e approverete il provvedimento in esame, ma abbiamo la consapevolezza che ci troveremo a dover ridiscutere seriamente di problematiche e di misure in campo di contenimento e risanamento dei conti pubblici e contenimento della spesa. Da questo punto di vista, voglio voglio dire, come punto di vista dell'opposizione e del Partito Democratico, che pensiamo non sia sufficiente un approccio ancora una volta di tipo minimalista.

che i carichi devono essere distribuiti in maniera relativamente equa. Questa manovra, pur essendo severa, dura, complicata per tutti, dovrà porsi l'ambizione di contrastare le diseguaglianze che stanno crescendo nel nostro Paese.

Il *welfare* va modernizzato, in Europa come in Italia, ma è un elemento fondamentale di tutela e di garanzia soprattutto per chi versa in condizioni di maggiore debolezza e difficoltà, dal punto di vista economico e sociale.

uno sforzo per valutare insieme, in uno spirito costruttivo, quali proposte e quale contributo offrire per predisporre un progetto che affronti in modo più organico e compiuto le esigenze e i problemi che ha il Paese, per darvi graduale soluzione.

credo che questo dibattito sia l'aperitivo di un dibattito molto più importante, legato al varo di una manovra che, evidentemente, dovrà mettere ulteriormente in sicurezza i conti pubblici

Ritengo che nei vari interventi dell'opposizione (riconoscendomi pienamente negli interventi dei relatori e nelle relative repliche, oltre che nei vari contributi di interesse della maggioranza),

di una difficoltà da parte dell'opposizione di trovare una linea che sia assolutamente unitaria, quanto piuttosto della difficoltà di interpretazione di un congiuntura che ha aspetti di complessità significativi.

Nasce da questa esigenza; un'esigenza maturata in un contesto di indicatori economici nazionali e internazionali che facevano intravedere in misura significativa un percorso di ripresa più forte rispetto ai dati che sono oggi alla nostra attenzione e che sono ricordati dagli operatori e dagli osservatori internazionali.

è chiaro che si deve comunque andare a razionalizzare l'intervento, che sappiamo non è stato esaustivo; ma non aveva la vocazione di risolvere i problemi della domanda e le difficoltà a fronte di una crisi così profonda,

che sotto certi aspetti si ricongiunge alle considerazioni del senatore Barbolini, ma sotto altri conferma una linea di correttezza del Governo che - ribadisco - dimostra questo cortocircuito complessivo. Il senatore Morando afferma sostanzialmente due cose:

ha; è discutibile che nella congiuntura in cui ci troviamo e nel momento in cui è stata presa questa decisione, sia corretto decidere di destinare spesa al sostegno della domanda.

che rappresentano la linea d'azione del Governo dei prossimi tempi. Quella era una fase in cui abbiamo ricercato risorse che il Paese sostanzialmente chiedeva - e ne chiedeva tante, ma ne abbiamo date di meno - con uno strumento che non andasse ad appesantire ed aumentare la pressione fiscale, che riprendesse un percorso di maggiore forza nei confronti della lotta all'evasione, ma che, allo stesso tempo, prevedesse una salvaguardia complessiva dei conti pubblici.

dobbiamo sempre cercare all'interno del nostro dibattito elementi che ci possano portare per forza in contraddizione ed in contrasto tra di noi. Noi abbiamo dei dati certi. Non dobbiamo farci del male in questa sede, nel momento in cui a livello internazionale ci viene riconosciuto

Dobbiamo evitare che questo elemento di possibile crisi sistemica si abbatta anche sull'Italia. Finora ci siamo riusciti, ma è opportuno metterci nelle condizioni di poter reggere bene per i prossimi mesi.

una scelta politica. Come destinare le risorse in modo produttivo a sostegno delle imprese, quindi al tema della ripresa, è argomento assolutamente serio, su cui il Governo è disponibile ad un confronto. Ha alcune idee e le espliciterà con una serie di interventi, ma è chiaro che gli argomenti sono sostanzialmente tre: come lanciare un percorso di aggancio allo sviluppo più forte rispetto a quello prospettato anche dagli indicatori internazionali e dagli orientamenti tendenziali; come sostenere in modo più efficace le imprese ed il nostro sistema produttivo; come fare attività di selezione sulla spesa pubblica. È chiaro che se si tratterà di un intervento comunque di

probabilmente riusciremo ad uscire da questa congiuntura più forti e con una capacità di crescita maggiore, ma se sbaglieremo questi passaggi ci sarà un danno. La possibilità del confronto sarà attorno a questi argomenti.

reciprocamente ci confermiamo la bontà delle scelte effettuate. C'è il tema del contenzioso, su cui c'è una posizione differente. L'Agenzia delle entrate ribadisce, al di là delle possibilità evocate rispetto a singoli casi, che è tema che non riguarda il Governo se non con una norma generale in cui abbiamo ribadito più volte che si tratta di un contenzioso che è difficilmente credibile nel tempo. Vista la lunghezza di queste procedure e soprattutto esiti che non hanno finora determinato entrate per le casse dello Stato, noi crediamo di essere stati efficaci da questo punto di vista, se è vero che abbiamo aumentato in misura significativa la capacità di far entrare risorse da parte dell'erario.

Quindi, il combinato disposto di ciò che riguarda tabacco, gioco, gli aggi ed altri aspetti di incasso che comunque vengono svolti dai nostri concessionari sul territorio, rappresenta un valore che che non è stato di riduzione, ma di crescita in questi due anni. La crescita determina ovviamente una serie di problemi problemi che stiamo cercando di affrontare. La crescita c'è stata perché, da una parte, il mercato è cresciuto; dall'altra è stata fatta - rivendico almeno questo - una buona manutenzione per recuperare fette di legalità in un mondo che per certi versi ha avuto ampi margini di illegalità fino ad oggi. Vi è molto da fare ancora nei prossimi tempi ed il potenziamento dell'amministrazione entra in questo tipo di logica, che non è solo il gioco ma è tutto ciò che riguarda il fronte incasso della nostra rete periferica. Questo argomento riguarda quindi la

dell'importanza di una rete sul territorio che resta vicino al cittadino e che consente di poter effettuare una serie di servizi. il tema della prevenzione rispetto alle dipendenze da gioco è serio. Ce ne faremo carico nei prossimi tempi: sta crescendo, il problema è oggettivo.

ed è giusto cominciare a lavorare. Il Governo se ne farà carico. Se ne parlerà ovviamente con chi ha deleghe specifiche dell'argomento, ma credo che non resterà lettera morta, poiché è alla nostra attenzione. Siamo altresì pronti ad affrontare in generale tutto questo tema con grande trasparenza,

abbia mantenuto la grande disponibilità, che ha dimostrato alla Camera. Mi rendo conto della lamentela che può esserci da parte dei senatori relativamente ai meccanismi determinanti dalla conversione di un decreto; la realtà è che il Governo si è presentato con grande disponibilità, tant'è vero che abbiamo modificato in misura significativa il decreto con emendamenti di carattere parlamentare, condivisi anche dal Governo e, se avessimo avuto margini di tempi interessanti anche in questa sede, ci sarebbe stata la disponibilità da parte nostra a ragionare su alcune di queste proposte, che avevano anche una ragionevolezza di fondo. Non abbiamo affrontato, tra gli altri argomenti, il tema delle cosiddette polizze dormienti, su cui vi è un problema che ribadisco in questa sede. Non si tratta di affrontare in generale un problema, su cui, riconosco, ci può essere un problema complessivo di equità sulla vicenda. Premesso che è stato un provvedimento straordinario, è chiaro che mettere mano all'aspetto dei diritti connessi a possibili ripristini

Quindi, il Governo non nega che possa essere un argomento da affrontare in tal senso. È altrettanto chiaro che nel momento in cui ci dobbiamo avvicinare ad un intervento significativo di compressione anche della spesa pubblica non è semplice pensare a forme di copertura che siano esaustive. Quindi, mi rendo conto che non risolviamo la questione; è in agenda e vedremo come affrontarla. In conclusione, signor Presidente, credo che questo sia complessivamente un provvedimento

545 miliardi per dare la scalata ad Antonveneta) e risponde: «Presidente, aspettiamo almeno che finisca il patto, il 18 aprile del 2005. Poi, a patto scaduto, mandiamo l'ispezione».

12 giorni dopo il primo *blitz* dei magistrati milanesi. Il presidente della CONSOB era la gola profonda di Fiorani, della procura e aggiustava le ispezioni. È uno scandalo e mi auguro che, affinché risulti